link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, onorevoli senatori, è venuto a mancare Giovanni Berlinguer, una figura eminente della Repubblica, uno dei migliori politici italiani, un servitore appassionato e competente delle istituzioni, dal Campidoglio alla Camera, al Senato, fino al Parlamento europeo. In ogni Assemblea ha lasciato un segno inconfondibile della sua presenza e anche in quest'Aula del Senato si ricordano i suoi contributi preziosi ed aperti al confronto con chi la pensava diversamente. Eppure, nel ricordarne il valore politico, mi pare di non aver detto quasi nulla sulla complessità e sulla ricchezza della sua personalità. Giovanni Berlinguer non è stato solo un politico, ma uno scienziato di ampi orizzonti, un militante dell'impegno sociale ed un intellettuale riconosciuto a livello internazionale. Sono impressionanti la vastità dei suoi interessi, la diversità dei campi di azione e la molteplicità dei linguaggi. A tenere insieme questa molteplicità di pensiero e di azione poteva essere solo una pregiata stoffa di umanità,

un piacere interloquire con lui, un'occasione imperdibile lavorare con lui ed un privilegio averlo come amico. Nei diversi gradi di relazione con lui rimaneva costante il suo stile lieve, generoso, semplice ed ironico. Non era privo di contrasti e, anzi, proprio da essi veniva il fascino della sua personalità, intransigente ed aperta, determinata e curiosa, solare e profonda. Alle radici di tutto questo, vi era la sua bontà: è davvero inusuale per un politico la parola «bontà». Questo carattere, quando viene ostentato, si capovolge nel fariseismo oppure si irrigidisce nella precettistica; quando invece viene dissimulato, agisce come una forza interiore che mette in movimento tutte le doti di una persona. In questo senso segreto, Giovanni era prima di tutto un uomo buono. Lo era perché amava la vita e a questo scopo intendeva piegare l'azione politica. La sua lezione è tutta qui: prendersi cura della relazione tra politica e vita. Quella relazione oggi rischia di essere recisa dalle algide tecnocrazie, dalle arroganze mediatiche, dagli inconsapevoli conformismi del nostro tempo. Il nesso tra politica e vita spiega la sua azione, prima di tutto come parlamentare. Il suo contributo è stato più intenso proprio nelle grandi leggi, che hanno suscitato un profondo coinvolgimento popolare: dalla legge sull'aborto, alla riforma psichiatrica, alla riforma sanitaria, di cui si ricorda una memorabile dichiarazione di voto, che svolse a nome del Partito Comunista Italiano. «La medicina è malata» si intitolava un suo libro, che negli anni Cinquanta anticipava, nella critica ai saperi correnti, i principi della riforma di vent'anni dopo: la prevenzione della salute, l'attenzione alle condizioni ambientali e lavorative, la lotta alla disuguaglianza nell'accesso alla cura. Sono questioni che ancora negli anni Duemila egli riteneva centrali, sottolineando da un lato i grandi progressi della scienza medica e allo stesso tempo il paradosso di un mondo diviso tra i problemi dell'obesità e quelli della morte per fame. Il primo suo libro che mi capitò tra le mani è stato «Borgate di Roma», scritto insieme a Piero Della Seta. L'impegno del politico, che si occupa della vita dei baraccati nella periferia della capitale, si intrecciava con la razionalità e la sensibilità del medico del popolo. Quel libro fu poi utilizzato contemporaneamente come libro di testo all'università, nella nascente disciplina della sociologia, e come manuale d'uso nelle sezioni di partito e nei comitati di quartiere. tra salute ed eguaglianza lo ha reso famoso nei Paesi latinoamericani, non solo a livello accademico, con l'ampio risalto dei suoi studi, ma anche per il riconoscimento popolare. ebbe a dire in un consesso internazionale: «Da noi Giovanni Berlinguer è una leggenda». Come è accaduto spesso a grandi italiani, gli capitò di essere conosciuto meglio all'estero che in patria. con il suo prestigio ha portato un contributo prezioso negli organismi internazionali, nell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e nello studio delle determinanti sociali della salute - come ha ricordato stamani il Presidente dell'apposita commissione dell'OMS, Michael Marmot,

nella quale contribuì a superare fratture ideologiche, proponendo una bioetica quotidiana, come autocoscienza della vita delle persone - e nel Parlamento europeo, con contributi decisivi per le risoluzioni sul cambiamento climatico. Giovanni Berlinguer è stato un innovatore in tutti i campi, anche nel suo partito. Nel PCI ha contribuito a superare le angustie ideologiche, volgendo sempre lo sguardo ai cambiamenti del mondo, spesso in anticipo rispetto agli altri dirigenti. È del 1973 una sua analisi su informatica e democrazia, che solo oggi, con l'avvento della rete Internet è diventata questione cruciale. Non ha mai avuto paura del nuovo, inteso come seria analisi del cambiamento. Divenne invece sospettoso, negli anni Duemila, del "nuovismo" come retorica, che rischia di nascondere il conformismo. Denunciò questo pericolo quando venne candidato alla segreteria dei Democratici di Sinistra, in un memorabile discorso, riprendendo un apologo di Rossini, che aveva giudicato il lavoro di un giovane compositore, dicendo: «Ciò che è bello non è nuovo e ciò che è nuovo non è bello». Giovanni si fermò lì: noi andammo avanti, fondando un nuovo partito, ma proprio per questo, ogni giorno, abbiamo il dovere di dimostrare che il nuovo è davvero bello e che della tradizione stiamo prendendo le virtù, lasciando indietro i difetti. Tra le virtù che Giovanni raccomandava c'era l'attenzione alla questione morale, riprendendo, senza mai ostentarla, l'eredità del fratello Enrico. Nella corruttela - diceva - la politica non solo compie un danno verso lo Stato e un'ingiustizia tra i cittadini, ma delegittima se stessa, perde la dignità e quindi la forza per cambiare le cose. Ma forse la ricchezza della persona si vede anche nelle sue attività più eccentriche, apparentemente minori. La relazione politica-vita era ricercata anche negli studi entomologici, che liberavano al massimo grado la sua curiosità: dallo studio sull'operosità delle api al mondo delle pulci - che, nella sua analisi, ha influito sulla storia, decidendo le sorti di grandi battaglie più che la genialità dei generali - fino a quella singolare usanza di tenere in casa un piccolo leopardo, cercando una dimensione domestica di quella vitalità apparentemente inquietante. La relazione tra i viventi era il suo assillo, ma una sorte amara lo ha colpito, lo ha segnato negli ultimi anni, proprio con la malattia che impedisce le relazioni con gli altri. Così, signor Presidente, ci ha lasciati Giovanni Berlinguer, in un mondo chiuso, senza parole. Se n'è andato poco dopo la scomparsa della sua amatissima Giuliana, come accade nei grandi amori tra due persone, dove nasce il bisogno di accompagnare l'altro non solo nella vita, ma anche nella morte. Negli ultimi tempi, quando incontrava gli amici, Giuliana diceva: «Venite a trovare il mio ragazzo!». Ad un amico che accettò l'invito, capitò la fortuna di essere riconosciuto da Giovanni e di ascoltare da lui una domanda incredibile: «Che cosa posso fare?». Questa domanda Giovanni lascia in eredità ai giovani: che cosa posso fare? Non solo per me, ma per noi, per la società, per il Paese. *(Vivi

voglio porgere, a nome dei senatori di Sinistra Ecologia e Libertà e di tutto il Gruppo Misto, la nostra vicinanza a Lidia, a Luisa, a Mario, a tutti i suoi nipoti. La scomparsa di Giovanni Berlinguer lascia un vuoto incolmabile non solo nella sinistra italiana, ma nel mondo della scienza e della cultura italiana. È un vuoto di quelli che impoveriscono il Paese, quando vengono a mancare quelle rare figure che sono state patrimonio di impegno e di concretezza, sempre alla ricerca di un bisogno ininterrotto di cambiamento. Era un medico e un professore universitario. È stato deputato, senatore, parlamentare europeo, presidente del Comitato nazionale di bioetica. È stato un ambientalista, un uomo mite e rigoroso, che non si inchinò mai alle sirene del compiacimento politico fine a se stesso. Dirigente del PCI, sempre attento a tutti i temi

del PCI fu candidato alternativo alla segreteria dei Democratici di Sinistra. In quell'occasione Giovanni Berlinguer, che raccolse il 34 per cento dei consensi, divenne, come molti ricordano, un importante riferimento per quanti, nel mondo della sinistra, non si riconoscevano in quella scelta prevalente. Nel maggio 2007, dopo lo scioglimento dei Democratici di Sinistra che porterà alla nascita del Partito Democratico, lascia il partito e fonda, e fonda, insieme con Mussi e molti altri, Sinistra Democratica, che darà vita, insieme a molti esponenti dei Verdi e del Movimento per la sinistra, a Sinistra Ecologia e Libertà. Ricordiamo con affetto la sua vicinanza ed il suo impegno, ad esempio, per la campagna elettorale per le europee del 2009. Ma Giovanni Berlinguer è stato negli anni Settanta - voglio qui ricordarlo - uno dei primi e dei pochissimi dirigenti comunisti, e più in generale della sinistra italiana, a mostrare interesse e attenzione per l'ecologia, tanto da essere tra i fondatori - pochi oggi lo ricordano - nel 1979 della Lega per l'ambiente. Lo ha fatto, come in ogni aspetto della sua attività politica, partendo dalla sua competenza e dalla sua professionalità. Lo ha fatto come uomo di medicina, indicando, denunciando e combattendo i danni enormi per la salute che comporta l'avvelenamento dell'aria e dell'acqua del nostro pianeta. Era un'epoca, bisogna ricordarlo, in cui nella sinistra italiana la sensibilità per questi temi e queste battaglie era scarsa, quasi inesistente. Prevaleva ancora una cultura strettamente industrialista, sviluppista, che tendeva a sottovalutare i danni della distruzione ambientale per tutti per i lavoratori. Il lavoro quotidiano e l'impegno di Giovanni Berlinguer sono stati da questo punto di vista davvero pionieristici. Fu proprio Giovanni Berlinguer a portare in Italia nel 1971, al famoso convegno dell'Istituto Gramsci su «Uomo, natura e società», Barry Commoner, uno dei padri fondatori dell'ecologismo scientifico mondiale. Fu proprio quel Commoner che, con i suoi continui viaggi in Italia, ebbe un ruolo decisivo nel gettare un ponte tra movimento ambientalista e movimento operaio.

del Partito Comunista come Fabio Mussi e i membri della sezione ambiente del PCI arrivano ad elaborare la posizione antinucleare che segnò il dibattito del 17° Congresso del Partito Comunista. In un suo importante libro su etica, scienza e salute, Giovanni Berlinguer sosteneva: «C'è un grande interesse per i casi che anticipano le frontiere future della scienza, ma si trascurano sempre più le implicazioni corali delle applicazioni scientifiche nella vita quotidiana. Da quando siamo in grado di agire su fenomeni vitali che dipendevano soltanto dalle leggi spontanee, e spesso a noi ostili all'evoluzione, gli interrogativi si sono infatti moltiplicati. La domanda principale non può essere: dove fermarsi; ma un'altra: dove orientiamo il nostro impegno. L'integrazione fra i diritti umani (e di tutti i viventi) e il progresso scientifico può costituire il fondamento di una bioetica laica, polemica verso integralismi e fondamentalismi, ma sensibile ai dilemmi posti che oggi nascono per ogni scienza». Questa è stata la sua ricerca in tutti questi anni. C'è un altro aspetto della personalità e del modo di intendere la politica di Giovanni Berlinguer che credo vada segnalato e valorizzato, tanto più in un momento come questo, quando i rischi di scollamento tra la società italiana e la politica, fra il Paese reale e la sua rappresentanza sono così forti. Giovanni Berlinguer era un politico nel senso pieno del termine, e tuttavia non divenne mai un professionista della politica, ma restò sempre un medico, che nella sua attività politica riversava la propria esperienza professionale e nella medicina, come nella ricerca scientifica, non perdeva però mai di vista i principi che ispiravano la sua militanza politica. E restò sempre uno scienziato, che coniugava la ricerca con il tentativo di mettere a punto una vera politica nazionale per la scienza, la ricerca e la critica continua della stessa scienza. Per Giovanni Berlinguer l'impegno nella medicina, all'università e nella politica non erano scindibili, erano facce della stessa medaglia. Così dovrebbe essere in generale per la politica. Così dovrà essere in futuro, se vogliamo ricostruire un rapporto solido tra la società e la politica. non erano mai astratte, mai dettate solo dall'appartenenza a un partito: discendevano direttamente dalla sua esperienza professionale, dalla sua esperienza umana. Fu così nell'impegno a favore dei più poveri, a favore dell'ambiente, nello schieramento appassionato a favore del Servizio sanitario pubblico, nello sforzo concreto per l'edificazione di una vera medicina sociale. Solo una politica di questo tipo, collegata all'esperienza diretta, immediatamente riconoscibile dai cittadini come espressione e rappresentanza delle loro necessità concrete e tuttavia profondamente radicate in un impegno politico non saltuario o superficiale, può ricreare quel nesso forte tra il popolo e i suoi rappresentanti che è venuto sempre più scemando negli ultimi decenni. C'è un ultimo aspetto della personalità di Giovanni Berlinguer che è necessario prendere a riferimento. Molti hanno ricordato il suo carattere, la sua mitezza, la sua disponibilità al dialogo con tutti. La sua politica era all'opposto di quella urlata che troppi, purtroppo,

aperta al dialogo e, tuttavia, ferma nella fedeltà ai principi e ai valori di fondo tornerà a essere credibile per i cittadini. È con questo che vogliamo salutare con grande affetto e rimpianto Giovanni Berlinguer.

Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo di Area Popolare, che mai hanno militato politicamente al suo fianco, si inchinano commossi alla memoria di Giovanni Berlinguer e sono grati al collega Tocci per l'elegante profilo politico che ne ha tracciato, compreso quel bellissimo accenno all'ultimo tragico destino di finire lui, medico e studioso della socialità del malato, proprio in quella tipologia di malattia che gli precludeva la socialità. Giovanni Berlinguer è stato parlamentare italiano in entrambi i rami del Parlamento. È stato parlamentare europeo e lo è stato sempre con straordinaria compostezza. Mi pare che il collega Tocci abbia usato l'aggettivo «mite» e la collega De Petris l'aggettivo «gentile». Forse aggiungerei qualcosa, se mi posso permettere di inserirmi nella tradizione storica e politica del mondo comunista. Non c'è dubbio che Giovanni Berlinguer appartenesse alla tradizione togliattiana, di quel Togliatti che, nella famosa intervista degli anni Cinquanta a «Nuovi Argomenti», sulla doppiezza aveva giustificato il parlamentarismo in funzione del leninismo e il leninismo in funzione del parlamentarismo. Giovanni Berlinguer è stato un parlamentare che non ha mai avuto una concezione strumentale del parlamentarismo. È stato un grande signore, anche quando era avversario implacabile di un Ministro della sanità di cui non condivideva la politica, ma nei confronti del quale non si è mai degradato a essere sciacallo. Da questo punto di vista, ogni riferimento al leninismo può non essere improprio nel caso di Enrico Berlinguer, ma è del tutto sbagliato nel caso di Giovanni Berlinguer. Basti una considerazione: Giovanni Berlinguer era un professore universitario, era uno studioso. Molte volte abbiamo visto colleghi di gran prestigio farsi prendere, se non in antipatia, in scarsa sintonia dai colleghi parlamentari per eccesso di piglio baronale o per eccesso, talvolta, di vanità dell'antipolitica, con il destino della banalità. Questo, in tante legislature, a Giovanni Berlinguer non è mai accaduto. Ha fatto il parlamentare di settore, di quel settore tra l'università, la scienza, la sanità e la malattia nelle sue implicazioni sociali

Ho avuto modo di conoscere così un avversario politico, sicuramente non un nemico; una persona corretta e coerente, un uomo di cultura, convinto delle sue tesi, che sapeva ascoltare e confrontarsi anche con avversari politici che sostenevano tesi a volte completamente differenti dalle sue.

IdV))*. Signor Presidente, nell'esternare a nome del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà la vicinanza alla famiglia, ma anche a tutti coloro che in politica hanno avuto la fortuna di accompagnare il percorso ed il cammino umano e di grande spessore politico di Giovanni Berlinguer, voglio in questa circostanza semplicemente ricordare alcuni momenti che ho avuto la possibilità di vivere al suo fianco, nel contesto delle istituzioni europee. È vero, Giovanni Berlinguer è stato un uomo politico con un pensiero politico molto distante dai miei convincimenti, ma nello stesso tempo ha avuto il merito di vivere con passione la posizione che la sinistra italiana è andata maturando rispetto all'idea di Europa in anni difficili, quelli cioè dell'implosione del sistema comunista e dell'evoluzione del pensiero della sinistra italiana sul tema dell'Europa.

che ha avuto il merito di tradurre in modo indelebile un suo profondo convincimento, che traspare anche in tutta la sua opera: mi riferisco all'antitesi profonda a quella concezione del potere per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. Per Giovanni Berlinguer l'uomo invece era tutto,

di fondo, su principi fondamentali, ma era invece una disputa quotidiana, era cioè la storia di tutte quelle persone che chiedevano che la politica aiutasse a guadagnare un po' più di senso alla vicenda di chi si trova di fronte al mistero della malattia e della morte, ci dà la misura della passione con la quale egli ha guardato all'attività politica e alla costruzione del rapporto tra politica e cittadini durante tutto l'arco della sua vita. È per questo che mi sento di unirmi doverosamente al cordoglio già espresso da tutti i colleghi. Sento come profondamente vere le parole espresse soprattutto dagli interventi dei colleghi Walter Tocci e Loredana De Petris, perché in tutta quella che è la grande storia e la vicenda della sinistra italiana è soprattutto la storia degli uomini a parlare, prima ancora che la storia delle idee. Dobbiamo tutti onorarci onorarci per avere conosciuto quest'uomo; soprattutto, dobbiamo sentire come un onore aver potuto vivere un pezzo della storia politica del Paese e delle istituzioni europee al suo fianco. *(Applausi).*

Credo che siano state sottolineate le sue qualità personali, il suo interesse per la persona, che gli derivava dal suo essere medico e fortemente cosciente dell'importanza sociale della sua professione e dell'importanza che hanno le politiche sociali rispetto alla generalità dei cittadini. In questo senso è bello che lo ricordino sia coloro che hanno appartenuto a formazioni politiche insieme a lui, sia coloro che sono stati, come noi, ben distanti dalle sue posizioni politiche.

divergenze tra coloro che vedono il bene comune in modo diverso, ma va riconosciuto lealmente, anche a chi appartiene a formazioni politiche diverse, che

lui l'ha fatto. Rendiamo omaggio a lui e uniamoci al cordoglio dei familiari.

la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 aprile. Oggi pomeriggio, dopo la conclusione della discussione generale sul disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, proseguirà l'esame del disegno di legge in materia di misure cautelari personali. Nella seduta antimeridiana di domani, che non prevede orario di chiusura, saranno esaminate la risoluzione della 14a Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo e le mozioni sul piano di razionalizzazione di Poste SpA, per le quali si è convenuto di procedere solo alle illustrazioni e alle dichiarazioni finali di voto. L'ordine del giorno prevede inoltre 1'esame della ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e le altre ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Nella seduta pomeridiana di *question time* il ministro Poletti risponderà a quesiti sui profili di attuazione della riforma del mercato del lavoro e sugli interventi in materia previdenziale. La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla mattina di martedì 14 aprile, con inizio alle ore 11, per la discussione del decreto-legge antiterrorismo e missioni internazionali. Il calendario prevede inoltre il seguito del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La seduta unica di giovedì 16 aprile, per la quale non è previsto orario di chiusura, sarà sospesa dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per consentire ai senatori di partecipare alla cerimonia celebrativa del 70° anniversario della Liberazione, che si terrà alle 11 presso 1'Aula della Camera dei deputati. Il calendario della settimana dal 21 al 23 aprile prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge sullo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative; il Documento di economia e finanza 2015, nonché il disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo. Nella seduta pomeridiana di giovedì 23 aprile avrà luogo il *question time*. Infine, nella settimana dal 28 al 30 aprile, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge collegato sulla semplificazione del settore agricolo, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nonché le mozioni sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti di animali e su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna. **Programma Signor Presidente, così come abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo, chiediamo che venga ascoltato in quest'Aula il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti, con delega al CIPE. Lo chiediamo perché, in ordine allo scandalo che sta coinvolgendo la CPL Concordia e altri, che ha evidenziato un ruolo molto forte di alcune cooperative in un sistema di corruttela molto diffuso, nelle varie informative si legge che l'attività di intercettazione in atto ha permesso di evidenziare la rete relazionale che Francesco Simone, *ex* responsabile responsabile relazioni esterne di CPL Concordia, è riuscito a creare nel corso del tempo, e che gli è funzionale a perseguire in tutti i modi i propri interessi. A tal riguardo, egli riesce ad avere un canale preferenziale anche con Luca Lotti. siccome il Sottosegretario ha la delega al CIPE, una delega molto pesante, noi chiediamo che egli venga a riferire in Aula in merito a questi fatti, e ci spieghi quali contatti esistono tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nonché segretario del CIPE, e questa persona che attualmente è in carcere. Quindi noi chiediamo che venga, per domani, calendarizzata la presenza in Aula del Sottosegretario, perché venga a spiegarci cosa sta succedendo.

Presidente, io non chiedo una modifica del calendario dei lavori, ma chiedo alla Presidenza di valutare (e chiedo anche agli altri Gruppi di esprimersi in tal senso, se lo ritengono opportuno)

di modifica del calendario con l'integrazione, nella giornata di domani, di un'informativa del sottosegretario Lotti,

Invito i colleghi che desiderano allontanarsi di farlo in fretta per consentire al collega Mazzoni di intervenire. il potenziale di crescita di un'economia può essere rafforzato anche da solide riforme strutturali, e la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni è certamente una di queste, anche se in questo testo non mancano certo le criticità. Peraltro l'*empasse* e il caos nell'attuazione del riordino delle Province gettano un'ombra anche sul cammino e sulla successiva applicazione della riforma Madia. L'Italia ha un'esigenza inderogabile: tagliare la spesa pubblica che continua ad aumentare in modo esponenziale. Tra il 2010 e il 2014 le uscite di parte corrente al netto degli interessi sul debito pubblico sono salite di più di 27 miliardi di euro. Nel 2014 la macchina pubblica è costata agli italiani circa 692 miliardi. Vale la pena ricordare, a questo proposito, che solo a seguito della riduzione delle unità di lavoro e del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici, introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi, in questi ultimi cinque anni la spesa per il personale è diminuita del 5 per cento. Dunque, è inutile girarci intorno: una seria riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni non deve prescindere dalla razionalizzazione della spesa pubblica, l'*ex* commissario alla *spending review* Cottarelli nel suo ultimo intervento, prima di tornare in America, non si è mostrato molto ottimista sui risultati di questa riforma, visto che gli obiettivi non sembrano includere, almeno non esplicitamente, il risparmio di risorse e - testuale - «non si può far finta che con i tagli non ci siano risparmi in termini di personale». In effetti, nel disegno di legge delega manca una definizione quantificata dei risparmi. O meglio, se va bene resta l'obiettivo di un 1 per cento annuale in meno sul totale della spesa. Ma dobbiamo chiederci quale spesa: quella pubblica complessiva - e saremmo a mezzo punto di PIL di spesa pubblica in meno - oppure un 1 per cento delle sole spese di funzionamento generale degli apparati della pubblica amministrazione, cosa che farebbe ridurre il risparmio a qualche centinaio di milioni l'anno? Il criterio pare sia demandato a decreti del Ministero dell'economia a sei mesi dall'approvazione della legge delega in Parlamento. Ma se questa riforma doveva essere il punto di partenza per fare finalmente un passo avanti serio nell'attuazione dei 30 miliardi di tagli previsti dal piano Cottarelli, allora siamo di fronte ad una falsa partenza. Il piano Cottarelli prevede, o meglio prevedeva una nuova disciplina dei licenziamenti individuali equiparabile a quella del settore privato. Ovvero, se il personale è in esubero in un particolare ufficio deve essere spostato altrove e chi si rifiuta di farlo cessa di essere in servizio. A Cottarelli va il merito non solo di aver previsto uno sfoltimento della spesa pubblica, ma pure di avere impostato una modifica importante nella gestione del pubblico impiego. Seguendo questo principio, il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che prevede la licenziabilità dei titolari dei nuovi contratti sia per ragioni economiche che per ragioni disciplinari, si dovrebbe applicare anche al pubblico impiego. Ma, ovviamente, vi è forte resistenza a questa norma da parte dei sindacati e il Governo si è adeguato, lasciando irrisolto il nodo di fondo e non applicando ai dipendenti pubblici le nuove regole del *jobs act*. Non c'è dubbio che il *jobs act* rappresenti uno dei temi più controversi insieme a quello della dirigenza pubblica, rispetto alla quale il Ministro punta sulla valutazione e la licenziabilità dei dirigenti inadeguati. Ebbene, in termini astratti, le linee generali indicate dal Ministro sembrano ineccepibili e condivisibili, quando dice di puntare su una dirigenza autonoma e indipendente dalla politica, alla quale si acceda per concorso e di volere meccanismi che, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della dirigenza, ne garantiscano la non inamovibilità, costituendo anche un presidio in più contro l'illegalità e contro la corruzione. Obiettivi giustissimi, ma siamo sicuri che vengano effettivamente centrati da questa riforma? La realtà è, invece, che in alcuni casi il disegno di legge finisce per cogliere obiettivi completamente opposti alle enunciazioni. Infatti, puntare su una sorta di abilitazione alla dirigenza, significa lasciare mano libera agli organi politici di assegnare gli incarichi con piena discrezionalità. Uno dei cardini della riforma è il cosiddetto ruolo unico nazionale di tutti i *manager* statali, insieme agli incarichi di durata triennale, rinnovabili una sola volta. Ma non va dimenticato un particolare importante, ossia che nella pubblica amministrazione ci sono sostanzialmente due categorie di dirigenti: quelli di ruolo, che hanno vinto un regolare concorso, e quelli nominati per contratto, che spesso sono cooptati negli enti locali dalla politica, seppur con incarichi a tempo determinato. Ebbene, con la riforma Madia i dirigenti di ruolo potranno un giorno trovarsi improvvisamente a spasso per mancanza di incarichi, pur avendo vinto un regolare concorso, mentre i *manager* nominati e cooptati dalla politica, che spesso hanno già un altro lavoro essendo di solito professori universitari, avvocati dello Stato o funzionari della stessa amministrazione che conferisce per contratto l'incarico dirigenziale, probabilmente potranno contare ancora sul salvagente degli agganci politici. Non va infatti dimenticato che il decreto-legge n. 90 del 2014 consente oggi agli enti locali di assumere *manager* cooptati senza concorso fino al 30 per cento degli organici, contro il 10 per cento previsto in precedenza. Per i dirigenti nominati, insomma, nei Comuni e nelle Regioni ci saranno ancora tanti posti a disposizione. Per chi ha vinto un regolare concorso, invece, c'è lo spettro del licenziamento. Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su un punto specifico: se vogliamo effettivamente riconoscere il merito, non si comprende per quale motivo la riforma diminuisca la parte della retribuzione legata al risultato, cioè quella con cui si premia chi concretamente raggiunge gli obiettivi. Infine, la riforma della pubblica amministrazione prevede l'abolizione della carica di segretario comunale e provinciale.

essendo di esclusiva scelta dei politici locali, che sono quindi liberi di determinarne criteri di nomina e compensi. Forse sarebbe stato più coerente individuare una figura più autonoma, sul modello dei segretari comunali come erano prima della riforma Bassanini. C'è stata, è vero, un'ampia condivisione tra i Gruppi politici sull'abolizione, tra tre anni, della figura del segretario comunale e provinciale, figura da sempre intesa come indispensabile per garantire lo svolgimento delle funzioni locali in autonomia e nel rispetto della legalità e a garanzia non tanto degli amministratori, quanto dei cittadini. E qui risalta proprio la funzione amministrativa rispetto a quella politica. In questo senso, la figura del direttore generale, che è stata uno dei principali fallimenti delle riforme Bassanini, configura una situazione di equilibrio precario perché posizionata tra politica e burocrazia, ognuna con le sue logiche, spesso in contrasto. questo vale, ovviamente, anche per la prevenzione dei fenomeni di corruzione negli enti locali. Per concludere, la catena di comando della pubblica amministrazione e la qualità del suo funzionamento risultano fondamentali, oltre che per fornire servizi efficienti ai cittadini, anche per organizzare la ritirata dello Stato in favore del mercato. Spero che nel corso dell'esame in Aula possano essere superate le criticità indicate, a partire dall'ex articolo 10 della riforma, che è a palese rischio di incostituzionalità.

Presidente, colleghi, questa riforma era stata annunciata per aprile, e ad aprile la discutiamo. Peccato che il riferimento fosse all'aprile del 2014 e non del 2015, ma conosciamo bene l'"annuncite" da prestazione del presidente Renzi, quindi direi che siamo nella norma. Un anno in più non sarebbe nulla se il risultato valesse l'attesa. Altro obiettivo nelle intenzioni del Presidente era riformare la pubblica amministrazione con il consenso dei cittadini. In effetti, il 30 aprile scorso, è stata lanciata l'OPA della grande consultazione pubblica, in pieno stile Renzi, *coram populo.* All'indirizzo *mail* del Ministero della funzione pubblica rivoluzione@governo.it (un nome, una garanzia) sono giunti oltre 39.000 messaggi. Che fine hanno fatto queste proposte? Dubito che i cittadini siano più ascoltati e considerati dei lori rappresentanti in Parlamento, ma magari il ministro Madia ha diligentemente integrato le proposte pervenute nella bozza di legge; magari ce lo farà sapere, sarebbe interessante. Per la buona scuola, la mia collega Blundo certifica che non sia accaduto. Entrando nel merito, la legge delega tocca tematiche importanti, sopratutto in materia di servizi al cittadino, procedimento e semplificazione amministrativa. Basta leggere i titoli per mettere tutti d'accordo su un cambio di rotta. Peccato, però, che siano principi già contenuti in altre norme mai applicate. Infatti, quante volte abbiamo già sentito parlare di interazione digitale tra cittadini e pubblica amministrazione? Mi riferisco all'accesso telematico, alle informazioni e ai documenti personali, ai pagamenti *on line*, al fascicolo sanitario elettronico e al superamento del cartaceo in genere, all'identità digitale. in tema di procedimento amministrativo, vi sembrano intuizioni originali la volontà di ridurre i passaggi, la loro durata, promuovere la digitalizzazione, aumentare la trasparenza? Queste belle e condivisibili intenzioni sono già sancite in disposizioni vigenti, quali la legge n. 241 del 1990, il decreto legislativo n. 82 del 2005, meglio noto come il codice digitale (modificato già due volte) nonché il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed altre ancora. Insomma, l'acqua calda già esiste. Come già esistono e sono attivi gli OIV (organismi indipendenti di valutazione) di brunettiana memoria, e con loro il sistema della premialità, degli incentivi e degli indici di *performance*. L'innovazione, oserei direi copernicana, sarebbe stata invece quella di trovare il modo per dare effettiva applicazione a queste leggi e magari in tempi ragionevolmente celeri e certi. In Italia, il problema non è produrre leggi; direi che ne abbiamo in sovrabbondanza. Dall'indagine conoscitiva effettuata recentemente dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui faccio parte, è emerso in maniera netta che il nostro ordinamento è caratterizzato da una stratificazione normativa, risultato dell'accumularsi di norme nel tempo, leggi ripetute spesso spesso senza il necessario raccordo con le norme previgenti. La Corte dei conti, il 20 novembre del 2014, mentre analizzava la stretta correlazione tra eccesso di leggi e corruzione, forniva un dato ormai noto: per abrogare una norma ne creiamo 1,2 nuove. Colleghi, riflettiamo. Il vero ostacolo, dunque, è rendere le norme esecutive. Per essere attuate, le leggi devono superare talmente tanti passaggi che nel frattempo si rischia di dimenticarsele e produrne di nuove. Sempre nell'indagine conoscitiva della Commissione semplificazione in materia amministrativa è emerso che in data 4 febbraio 2014 avevano trovato attuazione solo 405 degli 883 adempimenti previsti dalle leggi approvate durante il Governo Monti e solo 17 dei 394 adempimenti di di legge previsti dal Governo Letta. Non credo sia un azzardo pensare che tale *trend* prosegua invariato anche nel Governo Renzi. La causa? Il rinvio! Le norme approvate, cioè, non sono autoapplicative, ma per essere efficaci richiedono l'emanazione di atti ulteriori in tempistiche incerte. Senza considerare poi i concerti, le intese, le acquisizioni dei pareri, e chi più ne ha più ne metta (solo in questo provvedimento, ad occhio e croce, ne possiamo contare almeno una ventina). Insomma, la tecnica barocca e ridondante del rinvio è una delle principali cause della "mala-legislazione" e, di conseguenza, della "mala-amministrazione", che a sua volta si riverbera negativamente sia sulla libera iniziativa imprenditoriale, sia sulle disfunzioni ed i costi esagerati della pubblica amministrazione, sia sulla quotidianità dei cittadini, che ne rispondono con il loro tempo, risorsa non rinnovabile, economicamente in termini di qualità della vita e di salute, perché la burocrazia imperante non produce, ma logora e danneggia. In questa giungla normativa, diventa un'impresa individuare il corretto percorso da seguire per ottenere autorizzazioni, licenze e quant'altro permetta l'esercizio del diritto d'impresa secondo le regole, senza finire tra le fauci di Equitalia. I cittadini italiani lo sanno, ormai sono rassegnati; gli stranieri stentano a crederci e quando non scappano ci ridono sopra, come sta avvenendo all'Expo. la vera svolta sarebbe stata cambiare tecnica legislativa, ma questa legge ricalca e conferma la vecchia prassi. In conclusione, a questa legge manca principalmente un elemento fondamentale per determinare un autentico cambiamento del nostro sistema amministrativo: il coraggio di affrontare gli intoccabili del vero potere decisionale, la casta dei burocrati. Nessuna svolta, dunque, nessun cambio di rotta, nessuna rivoluzione, a dispetto dell'indirizzo di posta elettronica sfornato dall'ufficio *marketing* di Palazzo Chigi.

titanica - ed aver guidato il processo di modifica intensa e profonda portato avanti in Commissione, ma anche il Governo per la disponibilità a collaborare con la Commissione su temi così importanti. Sono tali perché riguardano un disegno di legge che, a mio avviso, ha l'ambizione di cambiare una delle leggi fondamentali dello Stato ed una visione dello Stato che poco per volta si affranca da quell'immagine

un ente totalmente sovraordinato rispetto ai cittadini, ad una nuova e moderna, in cui lo Stato ha un ruolo molto più affievolito, esiste una dimensione multinazionale europea e, di fatto, la sua funzione è quella di creare un *legal framework*, un contesto normativo nel quale si gioca il grande gioco delle relazioni economiche e civili tra i cittadini.

Esiste in un pluralismo normativo, all'interno dell'Unione europea, in base al quale non soltanto gli Stati, ma addirittura le grandi regioni industriali - per esempio la Baviera, la Ruhr, Lione, il Nord-Est italiano o Barcellona entrano in concorrenza fra loro, cioè diventano soggetti che fanno parte del grande gioco della concorrenza. Per questo è necessario che si costituisca una rete tra i servizi servizi burocratici, quelli amministrativi e la capacità di risposta del tessuto imprenditoriale di ciascun Paese e di ciascuna Regione. In un tempo in cui

un'iniziativa congiunta pubblico-privato. Il tema del *project financing*, che in Italia non è mai decollato, dimostra proprio come a fronte della disponibilità di iniziative imprenditoriali, sia mancata la capacità attrattiva dei territori di di rendere effettivi i progetti che erano stati ipotizzati. Di fatto il *project financing* si è risolto in un finanziamento di opere sostanzialmente di natura minore o di opere che hanno richiesto necessariamente un contributo significativo da parte dello Stato. Stato. Ciò non ha prodotto, però, quel volano per lo sviluppo del Paese che ci si attendeva. Oggi lavorare sui requisiti e sulle caratteristiche della pubblica amministrazione significa proprio cercare di intervenire su questo livello superare non soltanto la farraginosità della legislazione speciale, ad esempio quella che riguarda i progetti pubblico‑privati che prima ho richiamato, ma quella complessiva, nel quale si muove l'economia e la capacità imprenditoriale del Paese.

sicuramente caratterizzano molti livelli della nostra amministrazione, ma che sono in qualche modo scoraggiate da meccanismi, che vanno a penalizzare non soltanto il privato, ma anche il pubblico. Mi sembra dunque necessario valutare il disegno di legge in esame, non in base alla sua conformità a modelli astratti di natura ideologica, ma rispetto alla sua capacità di incidere in modo effettivo sulla realtà del nostro Paese.

la riforma dovrà essere ispirata a «principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi» e ai «principi di ragionevolezza e proporzionalità». L'introduzione nel nostro ordinamento di questi principi comporta dunque l'introduzione delle caratteristiche di semplificazione e di accelerazione dei servizi per i cittadini e le imprese, l'informatizzazione delle procedure nei pagamenti e nelle relazioni con i cittadini e le imprese, la riforma della conferenza dei servizi - che è sempre stato il collo di bottiglia bottiglia del processo decisionale della pubblica amministrazione - con l'adozione di un principio maggioritario, con la riduzione dei casi in cui è obbligatorio il parere della Conferenza dei servizi e con la previsione della possibilità di un esame anche asincrono e telematico dei documenti,

ha avuto, nei fatti, un'introduzione ancora parziale. Ricordo che in base a tale direttiva l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace, a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuti in debito conto i rischi e i pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. prevedeva anche che l'autorizzazione possa essere concessa non solo in base a una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita, derivante dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività, affinché quest'ultima sia legittima. Questi principi, insieme al principio della libera concorrenza dell'impresa, della libera prestazione dei servizi, dell'uguaglianza, dell'equità,

voto e un giudizio favorevole sui principi che sono stati indicati e, per questo motivo, non posso quindi che concludere esprimendo soddisfazione per il disegno di legge in Presidente, la ringrazio per l'attenzione, come ringrazio sicuramente il Ministro per l'attenzione che vorrà riservarmi. Vede, signora Ministro, io non farò un discorso d'ordine generale, ma concentrerò l'attenzione sull'articolo 7 del provvedimento, in particolare per le conseguenze che ne potranno derivare in materia di possibile ed eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in seno al Ministero dell'interno. Io considero questo aspetto non solo pericoloso, ma addirittura eversivo; e le spiegherò subito le motivazioni. Lei sa bene che il Corpo forestale dello Stato ha sempre trovato una propria collocazione nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari

Vede, il Corpo forestale dello Stato, come lei sa, è una polizia specializzata che si occupa del patrimonio agro‑forestale italiano, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, di salvaguardia della biodiversità, di prevenzione e repressione dei reati agroalimentari agroalimentari e ambientali, della protezione dei boschi dagli incendi e della salvaguardia del territorio. Esso ha una serie di compiti: la tutela dell'ecosistema attraverso attività di prevenzione e repressione delle violazioni, la tutela delle foreste e della biodiversità vegetale, la tutela della biodiversità animale, la sorveglianza delle aree naturali protette a tutela del patrimonio naturalistico nazionale, la protezione della fauna e della flora minacciate di estinzione, la tutela degli animali dai maltrattamenti, la tutela della fauna selvatica, lo svolgimento di attività di contrasto al commercio illegale di flora e fauna in via di estinzione ai sensi delle convenzioni internazionali, il contrasto del commercio di legno illegale, il monitoraggio e il controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto prevenzione e il contrasto di illeciti correlati al fenomeno degli incendi boschivi, il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, la tutela degli ecosistemi naturali attraverso attività di prevenzione e repressione di violazioni in danno di ambiente e paesaggio, l'esercizio di attribuzioni demandate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e derivanti da normativa comunitaria, lo svolgimento di attività di sorveglianza ed accertamento degli illeciti commessi in violazione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dal relativo danno e disastro ambientale, il controllo in ordine alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'attività agro-forestale. E qui mi fermo per brevità. Si tratta di tutta una serie di attribuzioni che afferiscono rigorosamente alle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che tra l'altro, anche dal punto di vista funzionale, hanno diretta attinenza con le *mission* del Ministero dell'ambiente e della tutela e del mare, da cui sussiste quindi una dipendenza funzionale anche per quanto riguarda la sorveglianza dei parchi nazionali, i rapporti per l'attività CITES e così via. queste attività non sono di fatto conciliabili con la *mission* del Dipartimento di pubblica sicurezza, del Ministero dell'interno. Quindi il mantenimento dei criteri elencati nella previsione normativa in questione non è conciliabile con l'assorbimento del Corpo nelle altre forze di polizia, in particolare nella Polizia di Stato. In particolare, se la riforma andasse a buon fine, non sarebbe possibile proseguire nella gestione sostenibile delle 150 riserve naturali statali oggi affidate al Corpo forestale dello Stato. Si verrebbero a creare sovrapposizioni territoriali delle articolazioni periferiche (Carabinieri e Polizia di Stato), che si troverebbero a gestire anche le 800, 900 stazioni già del Corpo forestale dello Stato; quindi sul territorio ci sarebbe una duplicazione di strutture, con relativo aggravio di spesa. Si genererebbero nuovi oneri, verrebbero meno le vigenti convenzioni del Corpo forestale dello Stato con le Regioni. Il paradosso di tutto questo è che vi siete anche contraddetti, perché, esprimendo parere favorevole in Commissione all'emendamento 7.117, di fatto noi avremmo la soppressione del Corpo forestale dello Stato in una situazione in cui permarrebbero i sei Corpi forestali delle Regioni e Province a statuto autonomo, con la possibile nuova istituzione, nelle altre 15 Regioni, di Corpi forestali regionali in aggiunta a quelli già esistenti presso le Regioni e le Province autonome. Come se ciò non bastasse, non dimentichiamo che nelle disciolte Province la polizia aveva, tra i compiti istituzionali, quello della sorveglianza ambientale. Si perderebbero, a causa di questo provvedimento, professionalità scientifiche e tecniche accumulate dai tre centri nazionali per la biodiversità in materia di salvaguardia del patrimonio genetico delle piante forestali autoctone, verrebbero meno competenze non si registrerebbero economie di spesa, non si riuscirebbe a portare avanti il monitoraggio, nel nostro Paese, del nostro patrimonio forestale in ottemperanza al protocollo di Kyoto e, cosa ben più grave, si darebbe libertà di movimento alle agropiraterie, alle agromafie che si occupano di traffico illecito dei rifiuti anche nel nostro Paese e si arrecherebbe conseguentemente un danno irreversibile all'economia nazionale, perché voglio ricordare che l'economia nazionale si basa anche sull'agroalimentare e su quel *made in Italy* che proprio quest'anno, in Expo 2015, noi vogliamo esaltare e vogliamo mostrare al resto del mondo. *(Applausi del senatore Albertini).* Mi pare quindi che questo sia un atteggiamento assolutamente contraddittorio e, come ho detto nella premessa E allora, fermiamoci prima che sia troppo tardi. Né la Polizia di Stato, né il Ministero dell'interno hanno alcuna competenza specifica per interventi di questo genere, mentre il Corpo forestale dello Stato ha alte professionalità che vengono riconosciute a livello europeo e a livello internazionale, che non potranno assolutamente essere pienamente integrate nel sistema di sicurezza nazionale.

che esistono sul territorio nazionale - mi riferisco alle vecchie polizie provinciali - e va fatto un discorso con le Regioni e con le Province autonome che hanno dei

la bellezza del nostro Paese, la sicurezza agroalimentare, il *made in Italy*, la lotta nei confronti di quelle perverse associazioni mafiose che hanno avvelenato e continuano ad avvelenare il nostro territorio, dalla terra dei fuochi alle altre decine, centinaia, migliaia di terre dei fuochi che sono

che ci separano dalla approvazione definitiva del provvedimento, almeno in quest'Aula, di valutare con grande attenzione cosa stiamo facendo. se si voglia andare su questa strada perché si sono sottovalutate queste argomentazioni o perché nel nostro Paese stanno prevalendo delle *lobby* industrialiste, delle *lobby* contro l'ambiente, delle *lobby* che alla fine non curano minimamente i reali interessi del nostro Paese. Paese. Proprio nell'anno della bellezza, proprio nell'anno dell'Expo, proprio nell'anno in cui dobbiamo dare al mondo la migliore immagine del nostro Paese, in cui dobbiamo essere capaci di vendere la bellezza del nostro Paese, ragioniamo su questi temi ed individuiamo quelle strade che possano garantire non la sopravvivenza di un corpo, ma come ho già detto l'interesse nazionale, che in questo caso significa salvaguardare la specificità del Corpo forestale dello Stato e le sue funzioni.

di voler fare. Addirittura gli diamo la delega a fare i criteri, che invece dovrebbero essere contenuti nella delega stessa. In molti punti di questo disegno di legge c'è scritto chiaramente

come facciamo a delegare la definizione dei criteri al Governo? Il disegno di legge nei suoi primi articoli interviene sulla Conferenza dei servizi, riducendo il più possibile il ricorso a questo strumento, cercando di velocizzare l'attività amministrativa. La logica è quella di velocizzare e non di ottimizzare, agendo sempre

un tema che ha visto coinvolti tanti, in questi anni, nel decidere tra un modello di polizie specializzate e un modello di polizia unica, suddivisa al suo interno in varie specializzazioni. Il dibattito è aperto e noi diciamo al Governo: «Fai tu. Decidi tu». Annulliamo tutto il dibattito che si è svolto in questi anni, e il Governo deciderà quello che vorrà. È una riga: riordino delle funzioni di polizia. A questo aggiungiamo l'abolizione del Corpo forestale. un senso di serenità: dopo aver ascoltato buona parte degli interventi, ho l'impressione che l'abolizione del Corpo forestale non dovrebbe passare. Dalla gran parte degli interventi che ho sentito, anche della maggioranza, sembra che siano tutti contrari all'abolizione del Corpo forestale (almeno quelli intervenuti e salvo qualche sporadico intervento).

Questa è l'unica cosa che viene detta in maniera chiara all'interno del riordino delle funzioni di polizia. Forse bisognava partire da carabinieri e polizia, che hanno funzioni sovrapponibili, anziché dal Corpo forestale.

abbiamo una legge delega in bianco. Sempre in questo provvedimento si legge dei dirigenti. Un emendamento è passato in Commissione. E devo dire che il testo uscito dalla Commissione, forse, in alcune parti è peggiorato rispetto alle volontà del Governo. Le andremo poi a vedere, emendamento per emendamento e articolo per articolo.

in mobilità (in aspettativa, spostato e poi ripreso) presso un privato senza alcun limite. Lasciamo al Governo la possibilità di definire ed ampliare le modalità di effettuazione della mobilità tra amministrazioni pubbliche verso il privato.

*(PD)*. Signor Presidente, egregio Ministro, egregio Sottosegretario, autorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a discutere e ad approvare la legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ci siamo più volte ripetuti, in sedi politiche ed istituzionali, che questo è un obiettivo centrale dell'azione del Governo Renzi. Questa profonda riforma del complesso della pubblica amministrazione potrebbe finalmente consegnare al Paese un'amministrazione pubblica più efficiente e più efficace, basata su meccanismi meritocratici. Potrebbe semplificare i servizi al cittadino e non ultimo, consentire di avviare quella staffetta generazionale che più volte è stata presentata agli italiani come uno dei principi di questa riforma. Vorrei intervenire proprio su questi elementi, facendo alcune considerazioni che, purtroppo, ad oggi non hanno trovato risposte operative e concrete nell'articolato che stiamo esaminando. L'11 novembre scorso ho depositato in Senato come primo firmatario, insieme ad altri colleghi, un'interrogazione in cui chiedevo di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo intendesse adottare per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, riconoscendo celermente diritti, ad oggi negati, a decine di migliaia di cittadini italiani vincitori di procedure selettive pubbliche nelle amministrazioni statali e negli enti locali. Abbiamo depositato questa interrogazione alla luce di alcuni dati straordinariamente allarmanti, sui quali ad oggi si evidenzia una sostanziale superficialità o, peggio, una incapacità di intervenire con strumenti risolutivi da parte delle amministrazioni locali. secondo il monitoraggio della funzione pubblica sugli enti pubblici locali e nazionali, sarebbero circa 4.000 in tutta Italia i vincitori di concorso pubblico e, quindi, coloro che vantano, secondo la giurisprudenza, un diritto soggettivo all'assunzione in attesa di quest'ultima. poi circa 80.000 gli idonei che, pur avendo superato tutte le prove concorsuali, non rientrano nei posti messi a concorso, ma che comunque possono godere, come in passato, del cosiddetto scorrimento delle graduatorie. I dati della funzione pubblica si accompagnano ad una riflessione politica del tutto evidente. In una fase in cui questo Governo ha saputo puntare tutto su una riforma del mercato del lavoro, introducendo meccanismi di tutela crescenti, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con l'obiettivo di favorire rapporti di lavoro sempre più stabili e duraturi, nonché di incentivare le imprese a nuove assunzioni, ci dobbiamo chiedere quale possa e quale debba essere il ruolo della pubblica amministrazione in tale ambito. Non è credibile una pubblica amministrazione nella quale i cittadini ripongono un legittimo affidamento nei procedimenti posti in essere dagli enti locali o, in generale, dall'amministrazione centrale dello Stato, e che poi manifesta una non capacità o una o una impossibilità, stanti le vigenti normative, a rendere operative quelle stesse procedure assunzionali dopo l'espletamento di selezioni pubbliche che, oltre a durare per diversi anni, con un aggravio di costi per l'Erario, non si concludono con le relative assunzioni dei vincitori. C'è, in tutta evidenza, una distonia fra quello che andiamo a riformare nel settore privato del mercato del lavoro, producendo opportunità e tutele, e quello che non riformiamo nel pubblico, dove ci sono imbarazzanti casi di procedure di selezione bandite nel 2010, concluse e per le quali non si è ancora proceduto ad una sola assunzione. Diretta conseguenza di questo ragionamento rimane l'aleatoria aspirazione ad una staffetta generazionale, che appunto non trova alcuna realizzazione pratica nemmeno nelle più benevoli intenzioni della riforma. Non troviamo, infatti, alcun meccanismo derogatorio che possa permettere a quegli enti, che si trovano nelle condizioni che ho prima menzionato, di poter procedere alle assunzioni derivanti da concorsi espletati e conclusi, sebbene durante la discussione e l'approvazione della legge di stabilità va dato atto al Ministro e al Sottosegretario di aver inserito una norma che doveva servire esattamente a questo procedimento, ma che purtroppo ad oggi non ha trovato alcuna attuazione.

mi rivolgo al Sottosegretario e al Ministro - come ad esempio quella in cui versa il Comune di Roma, nell'ambito del quale l'assorbimento, secondo i piani assunzionali presentati dall'amministrazione, di 1.995 vincitori di concorso pubblico (stiamo parlando di vincitori di concorso pubblico, e non di idonei che aspettano lo scorrimento della graduatoria), per 22 profili professionali (concorsi banditi nel 2010, secondo le norme che abbiamo approvato nel corso di questa legislatura), avverrebbe in almeno 15 anni a partire dall'anno in corso. dall'anno in corso. È una pubblica amministrazione che definisce le assunzioni di vincitori di concorso in tre lustri. Possiamo identificare queste procedure come rispondenti a quei principi di economicità, efficienza ed efficacia a cui dobbiamo e vogliamo ispirare questa riforma? Pongo l'attenzione del Governo su questi temi. Proprio per questo motivo intendo presentare un emendamento, che non vuole andare contro,

con molta abilità e capacità, il senatore Pagliari, che è un insigne giurista. Noi non riusciamo a spiegare ai vincitori di concorso come sia possibile che, quando un'amministrazione statale o comunale delibera un delibera un fabbisogno del personale - e quindi stabilisce quale sia il numero delle persone addette ai vari profili professionali, fa l'appostamento di bilancio, predisponendo i soldi per poter poi procedere all'assunzione,

È una prospettiva assolutamente reale che abbiamo il dovere, nelle more di questa riforma, di affrontare ed evitare. E sarebbe un grave errore se, parallelamente al *jobs act*, act*, non individuassimo misure puntuali e di rapida efficacia per risolvere questa problematica, che rappresenta un elemento centrale dell'impianto di legge di riforma che avete presentato all'attenzione del Parlamento.

ed è, nella realtà, la proiezione più tangibile e concreta che accompagna e caratterizza i termini astratti come "pubblico", "comune", "bene pubblico", "bene comune". Nella capacità di rendere tali sostantivi ed aggettivi come percepibili, e prossimi agli interessi dei cittadini, risiedono la volontà e la capacità di Governo. Pertanto, una riforma delle amministrazioni pubbliche, come quella di cui ci stiamo occupando oggi, potrà essere suscettibile di successo o di fallimenti nella misura in cui concorrerà, in maniera primaziale, a determinare vicinanza e coinvolgimento del *corpus* degli amministrati ad un progetto di generale visione, di crescita condivisa, di sviluppo sociale ed economico per tutti e per ciascuno. Viene in mente quel meraviglioso dipinto che è l'«Allegoria del buon governo» di Ambrogio Lorenzetti, anticipatore sul piano plastico, ben settecento anni fa, di un modello perseguito nei secoli, nelle varie età della storia dell'uomo, come ideale forma di organizzazione ed armonizzazione degli interessi individuali e collettivi, forse anche la ricerca della felicità in terra. Ricordiamoci che soltanto la Costituzione americana parla di ricerca della felicità affidata - come filosofia politica, come teoria e prassi - alla gestione della convivenza umana. La Costituzione della nostra Repubblica, invece, fondata sui valori della Resistenza, e quindi fortemente segnata da passaggi storici esperienziali, persegue obiettivi di civile convivenza, di armonizzazione delle diversità naturali e delle sovrastrutture sociali; parla di principi fondanti preordinati al pubblico bene ed al benessere degli individui e della collettività. Orbene, mettere mano alla riforma della pubblica amministrazione è come accingersi all'aratura stagionale di un vasto campo di principi, applicazioni, ambiti e comparti che, di certo, mostrano limiti ormai intollerabili, fortemente condizionanti, traumaticamente devianti del buon funzionamento dello Stato nella complessità delle sue forme, nei livelli di Governo territoriale e centrale. Tutti denunciamo le inefficienze. Tutti conveniamo sulla necessità di porre mano alla riforma. Ricordiamo altresì a noi stessi - giusto per sottolineare l'importanza dell'atto in oggetto evidenziato - che si deve al grande imperatore romano Adriano il paradigma moderno di funzione pubblica e di pubblica amministrazione. Teniamone conto quando, frettolosamente, archiviamo prassi e teorie che hanno finito per informare una cospicua serie di modalità gestionali universali. Lo vogliamo ricordare a questo Governo, lo vogliamo sottolineare alla sua maggioranza. L'Esecutivo Renzi e la coalizione di Governo non ritengano di dover ottenere una miriade di deleghe su temi, questioni e principi di cui il Parlamento è all'oscuro, di cui i cittadini saranno soggetti passivi, di cui l'ordinamento dello Stato (fatto di uomini e donne con facoltà di pensiero e di azione) non abbia preventiva informazione. È paradossale, infatti, che decenni di conquiste di diritti e di livelli di partecipazione - penso, ad esempio, agli organi collegiali nella scuola e nelle università - continuino ad essere mortificati dal fare muscolare di un Governo, sì motivato da finalità significative ma che nei fatti calpesta le dissonanze ed annulla la condivisione. Peccato, perché su importanti categorie del disegno di delega si potevano registrare le sensibilità più autentiche del Paese, le intenzioni più nobili della cittadinanza attiva. Nulla, infatti, è dato sapere su cosa realmente sarà fatto di conquiste basilari nel processo di semplificazione e snellimento come la Conferenza di servizi, l'istituto del silenzio-assenso, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la dirigenza pubblica; del perché vengano archiviate figure emblematiche degli enti locali qual è il segretario generale. A tale scopo non sarebbe stato più opportuno e confacente alle reali necessità di sindaci ed amministratori rivalutare e riqualificare questo ruolo di pubblico funzionario, responsabilizzandolo nell'ottica di dare legittimità agli atti prodotti dai Comuni ai fini della trasparenza e della lotta alla corruzione? Peccato che interi corpi di polizia vengano soppressi ed ancora non si conosce quale sarà la branca della pubblica sicurezza che che ne assorbirà le funzioni. Mi riferisco al Corpo forestale dello Stato, benemerito e vetusto di significative imprese, presente in zone montuose e rurali, lungo i fiumi e nelle aree protette, nei parchi naturalistici nazionali e regionali. I risparmi che si vogliono perseguire nella riorganizzazione delle forze di polizia, francamente troppe e necessariamente prive di mezzi, dovrebbero basarsi piuttosto sulla centralizzazione degli acquisti, sull'introduzione dei costi *standard* e nel e nel rinvigorimento dei commissariati alla spesa. Ma, ragionevolmente, lasciamo al loro posto i forestali, dotiamoli di tecnologie avanzate nella lotta al crimine ambientale. Contribuiranno a fare dell'Italia un Paese che rispetta il paesaggio e concorre alla valorizzazione delle risorse naturali e delle vestigia del passato, per creare nuova occupazione e imprenditorialità nei beni culturali ed ambientali. Siamo delusi dal modo di agire del Governo. Non c'è dubbio che tale modo di procedere risenta di impostazioni propagandistiche dell'Esecutivo che, in tempi di verità giustamente reclamate dalla popolazione ed ineludibili, piuttosto l'annuncio sensazionale, il *tweet* tempestivo e *tranchant* che non i fatti concreti: guadagnare con la riforma della pubblica amministrazione i titoloni dei quotidiani e rinviare a tempi successivi i provvedimenti attuativi. È accaduto con la legge di delega fiscale. È il caso di ricordare al Governo che il Paese è maturo, da sempre, per recepire gli effetti dell'aria nuova, a patto che sia aria pura, non contagiata dal virus della demagogia. *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro e rappresentanti del Governo, nella storia della Repubblica italiana l'ambizione di riformare la pubblica amministrazione è stata la più ricorrente, forse la più ostinatamente perseguita e, insieme, la più frustrata. Non è certo questa la sede per ricostruire le cause di questi parziali o totali fallimenti che - a mio avviso - in gran parte risiedono nel carattere di una riforma che, per essere davvero efficace, dovrebbe avere carattere sistemico, investire cioè, nello stesso momento, tutti gli aspetti del funzionamento delle amministrazioni (dal profilo culturale degli addetti all'organizzazione, dalle regole del procedimento ai controlli) e che, invece, ogni volta è inevitabilmente parziale, e per questo lascia pericolosi varchi in cui inevitabilmente si incuneano i sabotatori delle riforme. Dunque, la sfida che il Governo ha lanciato sulla pubblica amministrazione è forse la più coraggiosa ed anche la più rischiosa, perché la scommessa è di riuscire dove molti altri hanno fallito. Oggi, però - a mio avviso - ci sono due condizioni del tutto inedite che possono indurre ad un certo ottimismo circa l'esito finale della sfida. In primo luogo, l'attuazione del nuovo assetto amministrativo

In primo luogo, l'attuazione del nuovo assetto amministrativo sarà gestita da una nuova leva di alti dirigenti pubblici, dirigenti coinvolti in una grande operazione di rinnovamento e di investimento di fiducia nei loro confronti. Non vi è dubbio, infatti, che, negli ultimi venticinque anni, i vertici dei gabinetti e delle burocrazie ministeriali hanno regolarmente teso a sterilizzare, direi lobotomizzare, le innovazioni contenute nelle diverse riforme nella fase della loro attuazione. Oggi non dovrebbe più essere così. Il secondo fatto nuovo è che questa riforma si propone di puntare tutto - o almeno così dichiara - sulla transizione al digitale: una leva potente, che può far fare un salto di qualità all'intero sistema pubblico

dai Ministeri, un *manager* per la transizione al digitale. Si creerà in questo modo una sorta di *network* di *manager*, agenti del cambiamento la cui missione sarà guidare non solo l'innovazione tecnologica ma, in primo luogo, la riorganizzazione dei processi e, di conseguenza, delle strutture e degli uffici

negli ultimi decenni, quando alla valutazione sono stati ancorati meccanismi riformatori che, in effetti, sono rimasti di fatto inattuati perché l'intero sistema era costruito su qualità e merito legati alla valutazione. Oggi, la leva del digitale può consentire questa trasformazione sistemica. È un'opportunità storica ed imperdibile, che altri Paesi stanno già utilizzando e che, se non fosse colta in tutte le sue potenzialità, aggraverebbe ancora di più quell'*handicap* competitivo che rallenta la nostra economia. tuttavia, ciò che qui manca - lo ripeto - è la consapevolezza circa le implicazioni e l'impatto che la rivoluzione digitale avrà sull'organizzazione amministrativa. Nel disegno di legge sono previste disposizioni opportune e importanti, peraltro anche migliorate dalla Commissione, sulla Conferenza dei servizi, sul silenzio-assenso, sull'autotutela, sulla concentrazione e sul coordinamento delle attività di verifica, di ispezione e controllo; norme che puntano, giustamente, a dare certezza

come strumento non solo di partecipazione e di controllo delle attività pubbliche, ma anche come prima misura di prevenzione della corruzione. Peraltro, si tratta in alcuni casi di norme norme quasi integralmente già previste da leggi in vigore, ma rimaste inattuate perché hanno bisogno di gambe solide su cui camminare. Hanno bisogno, cioè, delle organizzazioni efficienti e di qualità del personale che vi opera. Sull'organizzazione, il disegno di legge contiene norme utili ed opportune, a cominciare da quelle che tendono a qualificare e rafforzare il ruolo di coordinamento legislativo ed amministrativo della Presidenza del Consiglio, per contrastare le azioni di interdizione e di ostruzionismo talvolta messe in atto dai singoli Ministeri, e molto spesso, in passato, all'origine anch'esse del rallentamento delle riforme (in passato, ma anche nel presente). sono, però, anche norme che sembrano riproporre - a mio avviso senza un'adeguata analisi critica - modelli di cui i fatti hanno già dimostrato la debolezza operativa. ad esempio, agli uffici territoriali del Governo, per i quali si rinuncia - io credo - a ricercare nuove modalità di coordinamento territoriale delle attività statali, magari sfruttando appieno il processo di digitalizzazione. Su altri temi che richiederebbero finalmente interventi chiari e netti c'è - mi permetto netti c'è - mi permetto di sottolineare - una eccessiva timidezza. Tra questi, il tema delle forze di polizia. Personalmente sono d'accordo, come credo molti altri colleghi, sulla prospettiva - speriamo, non è detto e non è scontato - di un nucleo specializzato di polizia ambientale al posto di un corpo *ad hoc*; un nucleo che, lungi dall'abbassare la guardia sui reati ambientali, al contrario la integri con indagini di con indagini di altissima specializzazione, perché riguardano organizzazioni internazionali, come le ecomafie, rispetto alle quali una polizia territoriale, come di fatto il punto nodale che il disegno di legge non affronta a sufficienza - a mio avviso - è quello più generale della specializzazione delle forze di polizia: chi fa che cosa. Oggi tutte fanno indagini di polizia giudiziaria, comprese le intercettazioni; tutte fanno il controllo del territorio, tutte fanno ordine pubblico e tutte perseguono i medesimi reati con effetti negativi sull'efficacia, sui costi e sul coordinamento operativo. Credo che l'attività istintivamente ed automaticamente difensiva dell'esistente, che molte forze di polizia mettono in atto

anche tecnologica, e il valore delle forze di polizia, la cui qualità ci viene riconosciuta anche a livello internazionale. Allo stesso modo, si è tornati un po' indietro sulle camere di commercio, delle quali, certo, quasi si dimezza il numero, ma si continua a mantenere l'ambiguità sull'ambito di operatività, sulla moltiplicazione delle società operative e su un'autoperpetuazione di un ceto para politico che, in verità, non fa onore alla nostra imprenditoria. Ad ogni modo, due sono i punti chiave - a mio avviso - meno convincenti, sui quali credo, da qui all'emanazione dei decreti delegati, sarà opportuno

sostanzialmente dalle norme una sorta di *spoil system* regolato e basato essenzialmente su valutazione e merito. È una impostazione giusta e condivisibile, ma mi domando: se e fino a quando questo meccanismo, e cioè la valutazione, non sarà operativo - e sappiamo dall'esperienza quanto sia difficile farlo funzionare - quali saranno i criteri e i modi con cui regolare e far funzionare in modo efficiente questa sorta di mercato virtuale della dirigenza pubblica, senza senza cadere in un sistema in cui prevalga la discrezionalità dell'organo politico? Sulle società pubbliche, poi, direi che forse le norme sono troppe; norme che, però, non chiariscono alcuni concetti chiave, che mi auguro, nel corso

per il mercato e nel mercato? Dall'altra parte, non si definisce invece in quali altri casi si può optare per il modello societario e a quali criteri pubblicistici deve corrispondere l'oggetto sociale: si possono produrre vini, olii, attività turistica e di promozione? Lì il perimetro va definito. Allo stesso modo quali devono essere i criteri per l'affidamento *in house*? Quali le soglie minime di efficienza ed economicità in termini di fatturato, numero di dipendenti e/o in rapporto al numero degli amministratori, livello di disavanzo e di debito, costi *standard* e prestazioni erogate? Pochi ma stringenti criteri che servirebbero a disboscare la giungla delle 8.000 resistentissime società regionali e locali e ad avvicinarsi all'obiettivo più volte indicato dal Governo. Credo che nel corso della discussione poche ma puntuali modifiche potrebbero aiutare il Governo a realizzare questo decisivo progetto di modernizzazione del Paese: a questo tenderanno le proposte emendative elaborate da me con alcuni colleghi, nell'intento di rendere più forte ed incisiva la riforma. Per questo, mi auguro potranno essere valutate positivamente dal relatore e dal Governo, che peraltro ringrazio per il lavoro di grande apertura, disponibilità e collaborazione svolto nel confronto in Commissione. IdV))*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, cari colleghe e colleghi, non cederò alla tentazione di affrontare quest'importante argomento dal punto di vista del senatore di opposizione che guarda in maniera critica qualunque cosa possa provenire dalla maggioranza e dal Governo. Mi sforzerò di affrontarlo, invece, dal punto di vista della sostanza, proprio perché un argomento come la riforma della pubblica amministrazione merita quel rispetto e quella capacità di dare un contributo richiesti a prescindere dall'appartenenza politica o dal raggruppamento all'interno dell'istituzione del Senato. Comincerò quindi con il dire che

di oggi, che mirano a migliorare il testo emerso dalla Commissione, dove in verità alcune proposte emendative da noi presentate sono già state accolte. Le riteniamo assolutamente essenziali, alcune riguardano proprio il tema della digitalizzazione e dell'ammodernamento informatico della struttura dello Stato, che è la vera riforma

la modifica del sistema delle camere di commercio. Non riusciamo ad intendere questa volontà pervicace dello Stato centrale

questi argomenti, tra l'altro, abbiamo assistito ad un dibattito piuttosto ricco, tanto che non si riusciva a distinguere chi fosse senatore della maggioranza e chi dell'opposizione. o, per lo meno, suggerimenti importanti, sono arrivati durante il dibattito da parte di tutti i settori del Parlamento. Questo indica un primo limite della scelta effettuata. Si è scelto

al riordino degli organi di polizia: non si può lasciare un argomento così importante per la vita quotidiana del cittadino italiano nell'ambito di una delega

Presidente, dovremmo poi andarci a fidare di un Governo, che più di un anno fa ha ricevuto una delega da parte del Parlamento per emanare i decreti fiscali. Dopo più di un anno, credo che lo stesso Governo, che oggi ci chiede l'approvazione di un'altra delega,

la mera potestà di decidere il bello e il cattivo tempo, il come e il quando, nella forma e nei contenuti: non è questo ciò che il Parlamento può consentire al Governo Renzi. Se mi consentite, non è questo che il Parlamento può consentire

di un'urgente e necessaria riforma della pubblica amministrazione, per il fallimento pieno di quella concezione - tutta figlia di una cultura, che purtroppo avete e perpetrate - che vede nella pubblica amministrazione

questa vostra visione è fuori dal mondo, fuori dal tempo e lontana dalle necessità e dalle urgenze che oggi vive il nostro Paese. Il cittadino oggi avrebbe bisogno di strutture e infrastrutture statali non solo più snelle e meno costose, ma soprattutto più rispondenti alle esigenze della propria quotidianità. Una piccola e media impresa italiana oggi vive sotto il controllo costante di tutte le autorità, non solo di polizia, ma anche di controllo amministrativo: se ne possono contare fino a 21 diverse

Ciò non comporta la naturale allergia nei confronti dei controlli rispetto alle proprie attività interne, ma comporta semplicemente il dispendio di energie, di forze, di ore lavoro e di ore di attività imprenditoriale, che vengono sottratte da uno Stato che non si dimostra amico dell'attività imprenditoriale e del cittadino, ma soltanto un Cerbero controllore. E non è così, non è questa la visione che abbiamo dello Stato Liuzzi poco fa citava esempi nobili della visione, che risalgono fino a settecento anni fa. Ma è una visione e un'impostazione che noi vorremmo fosse completamente diversa; che partisse da un punto di vista, da una prospettiva, da un angolo di lettura che non è il vostro e non è quello che state proponendo al Governo. Vediamo che pochi sforzi vengono messi in quella digitalizzazione che darebbe davvero uno *sprint* alle attività imprenditoriali e alla tranquillità della vita del cittadino, che potrebbe fruire dei servizi della pubblica amministrazione senza code interminabili o senza perdita di ore di lavoro. Avete una visione della dirigenza

mirate più alla regolarità delle strutture e delle infrastrutture. In questa fase del dibattito - credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione - voglio dire che guarderemo con attenzione all'atteggiamento

con lo spirito di ritenere che oggi è ineludibile il tempo della riforma della pubblica amministrazione; però è anche importante

Salutiamo il secondo gruppo delle studentesse e degli studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Magrini e Marchetti» di Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Benvenuti al Senato.

in primo luogo voglio cogliere questa occasione per dare atto al collega Pagliari, relatore di questo disegno di legge, del gran lavoro fatto, producendosi ed inducendo nel Governo, in generale piuttosto restio, alcuni rilevanti, ancorché sofferti, momenti di ascolto. Qualsiasi Governo che voglia accreditarsi come riformatore prova a mettere mano alla pubblica amministrazione. In effetti, quello di rendere efficiente la pubblica amministrazione e renderla quindi capace di svolgere il proprio compito al minor costo è la grande sfida di tutti i Governi che si sono succeduti in Italia. A dire il vero, oggi appare complicato anche renderla solo efficace, cioè capace di svolgere il proprio ruolo in modo soddisfacente, indipendentemente dai costi di produzione dei servizi. Eppure di tentativi di riforma non ne sono mancati, per lo più tesi dichiaratamente a distaccare le funzioni politiche di indirizzo da quelle amministrative di gestione e a rendere l'attività amministrativa trasparente verso l'utenza. Francamente, la sensazione che si trae da uno sguardo d'insieme è uno scenario desolato, in cui pochi successi effimeri e parziali stentano a mostrarsi in un magma di insuccessi più o meno riconosciuti. Di fronte a tanti infruttuosi tentativi di riforma, sorge il dubbio che le cause reali del malfunzionamento della pubblica amministrazione italiana non siano mai state realmente aggredite nel loro complesso e nel loro punto nodale e che i pochi successi si siano verificati in quei pochi casi in cui un soggetto politico abbia unito in sé incisività e voglia di far bene (binomio appunto raro, purtroppo). In effetti siamo convinti che le pubbliche amministrazioni italiane, così come sono, costituiscono il prodotto della politica italiana così com'è stata e, peggio, com'è diventata negli ultimi Per intenderci, i vecchi burocrati (non gli impiegati degli uffici, ma l'alta dirigenza) sono stati insediati dalla politica ed hanno messo radici e di quelle radici si sono serviti per negoziare con i politici sopravvenuti (sulla base del vecchio criterio per cui il politico passa ed il burocrate rimane). Fino a quando la politica ha deciso di distinguere il proprio potere di indirizzo da quello gestionale (senza rinunciare realmente al potere di gestione, attenzione) e allora ha teso a sottrarsi alle responsabilità personali delle scelte di gestione, mantenendo però stretto il proprio controllo sulla permanenza dei burocrati al loro posto. Se quello che ho appena detto è vero (e, vi prego di credere, che lo è) da questa rappresentazione sono assenti i cittadini, destinatari finali del servizio. Per quello che riguarda la partecipazione dei cittadini è interessante un fenomeno che ho avuto modo di rilevare personalmente nella mia esperienza professionale: nei corsi di aggiornamento sul diritto di accesso che seguivo da giovane impiegato pubblico, con mia grande sorpresa e disappunto l'aspetto che veniva trattato più puntualmente erano i limiti che potevano essere opposti alle richieste di accesso dei cittadini.

sopravvento della normativa sulla *privacy* (interpretata quasi sempre in modo molto estensivo) tali limiti si sono moltiplicati (nella valutazione di quanto sto dichiarando bisogna tenere nel debito conto la difficoltà di mantenere aggiornato il personale sul disposto di leggi che

A nostro avviso, quello che dovrebbe andare a modificarsi nelle pubbliche amministrazioni sarebbe quindi la permeabilità di queste ai bisogni legittimi degli utenti (primo tra tutti la conoscenza dei processi per un funzionale ed un pregnante controllo di legittimità quando non di legalità). Per ottenere questo obiettivo - nei fatti - bisognerebbe cambiare la cultura del personale delle pubbliche amministrazioni e a questo si arriva con una netta volontà politica e con un bel po' di tempo. Il tempo non è mancato, la volontà politica sì. Ma venendo a questa legge delega: questa legge effettivamente cambia verso? cambia verso? È la volta buona? Mi permetto di immaginare queste espressioni precedute dal cancelletto tipico degli *hashtag.* A dire il vero, la sensazione che si trae da questi articoli è che si sia proceduto un po' "alla renziana", in presenza delle suddette difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione, si sia deciso di tagliare i nodi, per cui se le pubbliche amministrazioni non partecipano alle Conferenze di servizi, o non danno il proprio parere i tempi definiti o se una Sovrintendenza si mette di traverso, si procede a maggioranza, oppure non potrà più parlare successivamente. Insomma si riducono i controlli della pubblica amministrazione, che viene vista come un ostacolo al libero fluire dell'iniziativa privata. E questo, devo dire purtroppo, con buona pace anche dell'ambiente, anche del patrimonio storico artistico e financo della salute dei cittadini (sono espressioni testualmente tratte dalla legge delega). In sostanza quindi, di fronte ad una amministrazione inefficace, capace anche di impiegare il ritardo per non rispondere, si va avanti senza risposte. Si controllerà poi. E così si sceglie di ridurre il compito delle amministrazioni pubbliche nella vita del Paese, di tagliarle; basta guardare al modo in cui si è trattata la riforma delle Camere di commercio: fissarne il numero massimo, come se l'incremento dell'efficienza non possa e non debba essere ottenuto incrementando la qualità dei servizi e non solo riducendo i costi delle unità di Camere di commercio esistenti. Così come basta guardare all'ipotesi di disciogliere il Corpo forestale dello Stato incorporandolo in altra forza di polizia, senza tenere conto delle opzioni possibili, cioè incorporare nel Corpo forestale dello Stato i corpi forestali regionali o le polizie provinciali. si tiene conto del fatto che nel Corpo forestale dello Stato esistono competenze particolari che necessariamente dovranno andare a competere con le altre competenze di cui sono saturi gli altri corpi delle Forze dell'ordine.

faire*, contrabbandata per modernità. Per cambiare realmente verso, le pubbliche amministrazioni si devono muovere su programmi di lavoro realistici, apprezzati dagli utenti interessati. Quante volte ho avuto modo di vedere progetti operativi per l'anno approvati a ottobre dell'anno di vigenza, con una sorta di *fictio iuris*, che non lasciava contento nessuno nella sostanza? Le carte però erano a posto.

Noi di Italia Lavori in Corso abbiamo presentato degli emendamenti per spostare in questo senso l'impianto complessivo di questa legge delega. Criticando non ci sottraiamo al confronto, sulle cose. Signora Presidente, signora Ministra, il disegno di legge sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione ha impegnato i lavori della Commissione affari costituzionali per un lungo periodo, anche per l'importanza dei contenuti, che rappresentano la terza gamba del progetto di riforma istituzionale del Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, accanto alle modifiche costituzionali e alla legge elettorale. Il disegno di legge è ambizioso, ma è quello di cui il Paese ha bisogno considerato che tutti riconosciamo le disfunzioni di funzionamento della pubblica amministrazione. Contiene diverse deleghe di cui, alcune multiple, ma necessarie perché nessun Parlamento al mondo riuscirebbe a regolare nei particolari il complesso delle regole dell'assetto amministrativo. Tocca molte materie, dall'organizzazione dello Stato e delle forze di polizia, all'attuale dirigenza, dai segretari comunali alle camere di commercio, al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie. La *ratio* del disegno di legge è ottimizzare la produttività del lavoro pubblico rendendone più moderna l'organizzazione. A tal fine si prevede la carta della cittadinanza digitale e la Conferenza dei servizi, la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli *standard* di qualità. la valorizzazione del merito ed il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; l'introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali. I cittadini avvertono la necessità di cambiare, di liberare il Paese da molti condizionamenti ed arretratezze, l'avvertono in maniera più forte ed anche razionale, di quanto non capiti alle rappresentanze corporative e politiche. Come ho già esposto, quella che stiamo discutendo possiamo definirla a pieno titolo una riforma istituzionale, perché quella della pubblica amministrazione è una sfida su cui, in un Paese democratico e moderno, maggioranza e opposizione si confrontano con obiettività, entrando nel merito in modo costruttivo, ed è quello che correttamente è avvenuto in Commissione, grazie anche all'impegno del relatore, senatore Pagliari, collega, e che, mi auguro, avverrà anche in quest'Aula. La pubblica amministrazione non è né di centro né di destra né di sinistra. La pubblica amministrazione ha bisogno di rigore ed efficienza. Serve ad aiutare coloro che i servizi non possono pagarseli di tasca propria, serve ad aiutare i più deboli, serve ad aiutare i più poveri ed è su questi punti che si realizza nella società il contratto sociale. I cittadini pagano le tasse e devono ricevere in cambio dei servizi da una pubblica amministrazione seria, onesta, efficiente, che ha al suo interno il criterio della meritocrazia e della premialità. L'obiettivo è quello di combattere le clientele, gli sprechi, i costi, le inefficienze, fare quello che in tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi occidentali e moderni è la norma. Dobbiamo mettere i dipendenti pubblici nelle condizioni di essere motivati: il dipendente che lavora tanto e che guadagna quanto quello che lavora poco è un dipendente demotivato e invece, ancora oggi, le persone valide, quelle che sono davvero preparate e danno il massimo, non ricevono riconoscimenti. I dipendenti della pubblica amministrazione nel loro complesso, infatti, sono stati visti come la palla al piede dello sviluppo, come una casta autoreferenziale che s'impone come l'unico vero cliente della pubblica amministrazione. In realtà la maggior parte sono lavoratori che patiscono il non essere gestiti o l'essere gestiti male e rappresentano una grande opportunità per il Paese. L'industria più importante d'Italia è la pubblica amministrazione: dà lavoro a circa 3.300.000 persone, con un costo di 158 miliardi di euro all'anno, una cifra pari all'11 per cento del PIL. Sul fronte della qualità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, il principale indicatore disponibile prodotto dalla Banca mondiale nell'ambito del rapporto «Doing Business» colloca quest'anno il nostro Paese al 56° posto su 189, con un peggioramento di quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Con significative variazioni di produttività ed efficienza, si potrebbero ottenere insperati punti percentuali di incremento del PIL, che nell'attuale fase del ciclo economico difficile rappresenterebbe un dato di straordinaria importanza: l'amministrazione pubblica, dunque, da palla al piede a motore dell'economia italiana. Le risorse umane sono una potenzialità sostanzialmente mai gestita. La pubblica amministrazione ha sempre fatto mera gestione burocratica del personale ed ha trascurato, anche per colpa di un sindacato e di una politica distratti, l'adozione di tecniche tipiche del Governo e della valorizzazione delle risorse umane. C'è da arrabbiarsi quando si mettono a confronto gli imponenti investimenti fatti in formazione, ai quali non è seguito un incremento di produttività, determinando una spesa inutile e spesso, quindi, uno spreco. Si deve introdurre la rotazione degli incarichi «delicati», oggetto privilegiato delle lusinghe dei corruttori. In questi anni c'è stata la tutela dell'inamovibilità del pubblico impiegato, che ha reso difficile spostarlo perfino da un ufficio all'altro all'interno di uno stesso palazzo: una logica che rischia di apparire prevalente perfino rispetto ai valori della trasparenza e dell'indipendenza. La rotazione è un principio di garanzia, evita le incrostazioni in cui nasce il malaffare. Deve quindi essere chiaro a tutti che il tema del funzionamento della pubblica amministrazione è decisivo per la vita del nostro Paese: se essa funziona male, il Paese funziona male. Ciò può realizzarsi solo se la pubblica amministrazione reagisce ai due grandi fattori di crisi di cui soffre storicamente, ovvero un *deficit* di efficienza ed un *deficit* di legalità. La domanda di fondo della società è quella di avere una pubblica amministrazione più efficiente e più legale: non è possibile definire efficiente un'amministrazione non rispettosa della legalità, così come perde valore un'amministrazione formalmente e burocraticamente ineccepibile, ma inefficiente. La corruzione passa inevitabilmente dai suoi uffici ed è alimentata dalla cattiva burocrazia. È proprio su questo fronte che si gioca la battaglia per la legalità. Il concetto di pubblica amministrazione è ormai associato al male, all'errore, alla paralisi, ma in realtà incarna un'istituzione virtuosa, che è vitale in ogni Paese moderno. Purtroppo oggi ne sperimentiamo soltanto la degenerazione, quando è mala burocrazia, che si trasforma in un potere strisciante, basato sulla gestione delle pratiche e che fa della lentezza uno strumento per imporre la sua autorità. tuttavia cedere alle semplificazioni e pensare che tutti i dipendenti pubblici siano dei fannulloni. La giusta richiesta di un fisco più giusto, di un cittadino meglio servito, di una sanità più efficiente, di una scuola più moderna non potrà trovare risposta, se la macchina del fisco, dei servizi pubblici, della sanità, della scuola ha strutture arcaiche, procedure lente, personale scelto male e poco motivato. Il Governo, il Parlamento e la stessa pubblica amministrazione debbono ricordare, come amava dire Filippo Turati, che le tranvie non stanno lì per dare lavoro ai tranvieri, ma per trasportare la gente. In altre parole, l'obiettivo da perseguire è quello di fornire un miglior servizio ai cittadini, non di accettare gli interessi degli addetti ai lavori. Conoscendo e valutando, governando ed innovando, si supereranno i tanti problemi e le tante arretratezze che ho sottolineato. Il corretto ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione è essenziale per combattere la corruzione, contro la quale, oltre ai rimedi repressivi di natura penale, sostanziale e processuale, di cui abbiamo dibattuto con il disegno di legge anticorruzione, è forse più importante l'aspetto della prevenzione. Altri Paesi hanno concentrato l'attenzione proprio su quella e gli strumenti che utilizzano sono i codici etici, la responsabilità organizzativa, modelli di mappatura del rischio, procedure di controllo per verificare l'adozione di misure di salvaguardia. È la strada giusta, ma la prevenzione deve essere soprattutto cultura della legalità; c'è bisogno di una mobilitazione culturale che parta dalle scuole. È necessario ridare ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e fare loro capire che la corruzione si può combattere. La corruzione è un grande *iceberg*, del quale conosciamo solo la parte che viene scoperta; quella che ci interessa, invece, è quella che sta sotto il pelo dell'acqua, quella che non si vede, quella che non è ancora scoperta, quella che è di difficile stima. La corruzione è una tassa immorale ed occulta, pagata con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini, che erode e frena il prodotto interno e che dobbiamo tutti insieme combattere. In questa direzione è necessaria una legislazione degli appalti più chiara, semplice, trasparente, ed il superamento della stessa legge obiettivo che non ha prodotto i risultati sperati in termini dì realizzazione delle opere, ma anche sul piano della legalità. Quel che è importante è non illudersi che la minaccia di manette facili, la moltiplicazione di controllori e controlli e lunghi processi penali siano senza controindicazioni e per di più risolutivi. Come diceva Tacito: *corruptissima re publica plurimae leges*. Ci sono troppe leggi e sono poco chiare; sono uno strumento potente, ma il nostro sistema ne abusa perché con esse vuole regolare qualunque situazione creando più problemi di quanto ne risolva finendo così per paralizzare tutto, anche perché molte di queste leggi devono poi essere concretizzate da regolamenti operativi che nessuno emette e così restano inapplicate. credo di poter dire che con l'intervento legislativo in discussione ci si rivolge da un lato ai dipendenti pubblici cui è giusto restituire orgoglio per la funzione e dignità per la posizione, dall'altro ai cittadini tutti ed al sistema produttivo, cui non si può continuare ad imporre una pubblica amministrazione senza controlli di efficienza e qualità. Si vuole un'Italia migliore in cui i dipendenti pubblici non sono burocrati fannulloni, ma risorse per gestire uffici più efficienti in cui il merito sia premiato, chiedendo agli imprenditori di collaborare per rendere la legalità conveniente e alla politica di impegnarsi concretamente per dare soluzione ai problemi ed essere d'esempio ai cittadini. La semplificazione amministrativa e quella legislativa non sono solo un processo tecnico, ma soprattutto un atto politico. I Governi che si sono succeduti, anche se hanno tentato, non hanno avuto la forza ed il coraggio di compierla perché è costosa in termine di consenso. Valgono per il nostro Stato le parole di Tocqueville: «Il gusto per gli incarichi pubblici ed il desiderio di essere mantenuti dalle imposte non è da noi una malattia peculiare di un particolare partito, è la grande permanente infermità della nazione stessa». È un dovere fare questa riforma: lo dobbiamo agli italiani che, con la loro fatica ed i loro soldi, reggono il Paese e finanziano lo Stato; lo dobbiamo a coloro che ne hanno bisogno, a coloro che non ne approfittano e preferiscono essere seri ed onesti piuttosto che furbi. L'obiettivo condiviso da tutti è che la pubblica amministrazione torni ad essere un fattore di crescita del Paese e non un ostacolo. Come sostenuto dal governatore della Banca d'Italia Visco, legalità, buona legislazione, regolazione efficace delle attività economiche, pubblica amministrazione efficiente sono le principali componenti di un sistema istituzionale in grado di favorire innovazione e imprenditorialità e rimuovere rendite di posizione e restrizioni alla concorrenza. Ai cittadini toccherà il compito di distinguere il grano dalla malerba, impedendo ai parassiti di arricchirsi con le risorse indispensabili per lo sviluppo di un Paese, quelle che servono perché domani i nostri figli diventino protagonisti di un'Italia che sta già migliorando, nella quale sarà bello crescere e lavorare a testa alta sicuri dei propri diritti. *(Applausi

consentiva di affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, consentendo la gestione *in house* solo ove ricorressero situazioni del tutto eccezionali, che non permettessero un efficace e utile ricorso al mercato; che la tariffa del servizio idrico dovesse includere anche la remunerazione del capitale investito dal gestore. ha dato uno *stop* che doveva essere definitivo a questo schema. Sulla gestione idrica non si doveva più fare lucro. Anzi, andavano fermate le privatizzazioni e avviato un percorso di ripubblicizzazione. Erano obiettivi pienamente legittimi, che recepiscono molti principi della nostra Costituzione e non ledono le direttive europee. In seguito a specifica petizione popolare, le istituzioni europee hanno chiarito che questa è materia affidata ai singoli Stati membri. Erano anche obiettivi condivisi da una imponente galassia di movimenti, associazioni, comitati, consigli comunali e provinciali, ma anche da sindacati come la CGIL, da circoli come l'ARCI, da tantissimi elettori del Partito Democratico, che obbligarono ad invertire le proprie posizioni i loro stessi dirigenti, sempre che i dirigenti del Partito Democratico siano gli stessi. Non mi riferisco a Matteo Renzi, ma all'ondivago Bersani, prima favorevole alla privatizzazione dell'acqua, poi favorevole al *referendum* e, infine, elusivo e impalpabile. Ecco perché il *referendum* popolare è rimasto tradito, con atroci beffe peraltro. A Padova, prima del *referendum*, la quota non dovuta in bolletta era il 15 per cento. Dopo il *referendum*, a distanza di un anno, era salita al 17 Questo disegno di legge doveva, e deve, essere l'occasione per ridare dignità alla volontà popolare, mettere una parola di chiarezza sui servizi essenziali risolvere il mostro giuridico delle partecipate. Queste sono società che possono assumere raccomandati in elusione del Patto di stabilità. Ma tanto scaricano in bolletta i costi di un servizio che gestiscono in monopolio. Serviva rompere questo paradigma per cui privato sarebbe bello. Lo ha rotto il sindaco di Parigi, realizzando risparmi enormi dopo avere ripubblicizzato l'acquedotto. E invece nel testo del Governo compare tutt'altro perché deve essere chiaro che il testo dell'articolo 14 è il testo del Governo, rimaneggiato dal relatore secondo la volontà del Governo e votato in Commissione dalla maggioranza di Governo, per partito preso o per maggioranza presa si potrebbe dire. Questo disegno di legge è una tragica velina che il Governo ha scritto e passato al Parlamento. Dentro ci sono gli ordini che il Governo pretende di ricevere da noi. E noi dovremmo anche far finta di decidere.

quale comune, azionista di una società, preferirebbe una concorrente per un affidamento, con il rischio di vedere sterilizzato il valore delle azioni e perdere un bacino clientelare faticosamente costruito. Tutt'altro serviva. Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti: perché si prendesse un impegno a ripubblicizzare la gestione di inceneritori e acquedotti; perché almeno si lasciasse questa responsabilità alle amministrazioni locali; perché si prevedesse l'obbligatoria consultazione popolare su scelte di questa portata: niente, nemmeno per gli acquedotti comunali dei piccoli comuni montani. II Governo chiede mani libere par fare carne di porco del *referendum* popolare. E usa un testo camaleontico per ingannarci. Dice: «in base ai principi dell'Unione europea e tenendo conto del *referendum* 2011». In base ai principi dell'Unione europea che sul tema riconosce l'autonomia degli Stati?

Abbiamo chiesto che si scrivesse «nel rispetto del *referendum*», ma anche questo è stato rifiutato; anzi, in un'altra parte del testo sono previsti incentivi e premi per quegli enti locali che favoriranno la perdita del controllo pubblico dei servizi locali. E allora voglio raccontarvi quello che è successo a Padova per mano del sindaco Flavio Zanonato. a tutti i costi la municipalizzata che, insieme al Comune di Trieste, gestiva il servizio idrico e la raccolta rifiuti con il più grande inceneritore del Veneto. Regalò la gallina dalle uova d'oro alla società Era, guidata dal patto di sindacato dei comuni rossi dell'Emilia-Romagna, e non chiese di valorizzare le sinergie. È come se vendessi una moneta d'argento, proprietà dei cittadini,

È danno erariale? Lo sta accertando la Corte dei conti, a cui abbiamo presentato un esposto. Quello che è certo è che noi padovani, avendo perso il controllo, respiriamo quello che la società Era, grazie allo sblocca Italia, farà arrivare da ogni dove per essere bruciato a mille e cinquecento metri dal centro storico; mentre dai bilanci di Era ricaviamo che nel concambio non ci hanno dato nemmeno il valore del metallo. Del resto Zanonato fu ritenuto troppo sprovveduto dai magistrati per rendersi conto che trasportava mazzette ai tempi di Tangentopoli, ma tanto capace, dai DS prima e dal Partito Democratico poi, che lo vollero prima sindaco, poi Ministro, ora europarlamentare. A noi raccontarono che al Comune sarebbero arrivati succosi dividendi. Ma cosa sono i dividendi? Sono quello che rimane - lo spiego ai cittadini che ci ascoltano - dopo aver dopo aver pagato le spese e messo da parte gli investimenti. Sono soldi che vanno restituiti ai cittadini, agli utenti, altrimenti a casa mia si chiama «fare la cresta». E se la società è a capitale misto, con un 40 per cento di privati, per ogni sei euro che vanno al Comune, quattro arricchiscono quei privati. Non si può sopportare. Le ipocrisie affiorano come i teschi da una fossa comune. Durante la campagna referendaria il fronte del «no» diceva che solo la gestione sarebbe stata privatizzata. un emendamento, ad escludere almeno la privatizzazione, ancorché parziale, delle reti. E anche questo è stato bocciato. Del resto, da un Governo che si accinge a svendere le torri di trasmissione RAI a Mediaset, che cosa ci possiamo aspettare? I nostri emendamenti ora sono in Aula. Potrete respingerli ancora, ma questa volta lo farete sotto gli occhi di chi vi ha votato.

siamo chiamati oggi ad esaminare uno dei provvedimenti più importanti, ed al contempo più complessi ed ambiziosi, dell'intera legislatura. Nel corso della sua relazione, tenuta in quest'Aula qualche giorno fa, il collega Pagliari ha richiamato un paradosso ricorrente: come si può pretendere di riformare, con esito positivo peraltro, la macchina amministrativa italiana, se in questa impresa si sono già cimentati tanti illustri predecessori? Come si può pensare di riuscire a conseguire i risultati che neppure i maggiori esperti - ad esempio Massimo Severo Giannini, il più illustre amministrativista italiano del dopoguerra - sono riusciti a conseguire? La domanda è sicuramente legittima. La riforma della pubblica amministrazione, ne siamo pienamente consapevoli, non è cosa semplice, eppure è necessario intervenire per tentare di rende più snella ed efficiente la nostra burocrazia. Varie sono le ragioni che inducono a questa riflessione. Innanzitutto, è indispensabile eliminare gli sprechi e ridurre le inefficienze, ritengo, al fine di rendere effettivo

intesa come attitudine a conseguire efficacemente i risultati mediante un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. È solo con una riforma della pubblica amministrazione che tenda a rendere la sua azione aderente alle famose «tre e» che è possibile giungere ad un significativo taglio della spesa pubblica superflua di cui tutti che permetterà di conseguire non soltanto l'avanzo primario di bilancio, ma addirittura una graduale riduzione del debito pubblico e ancora, sicuramente, la riduzione del carico fiscale che grava su imprese e famiglie, per favorire in tal modo una ripresa dei consumi e un conseguente incremento del prodotto interno lordo. Risulterebbe, tuttavia, poco lungimirante e del tutto pericolosa un'operazione che tendesse a perseguire questi obiettivi riducendo i servizi offerti ai cittadini: la riduzione della spesa pubblica si tradurrebbe così soltanto in un decremento dei servizi a scapito della collettività e inciderebbe gravemente sugli *standard* sinora assicurati alla popolazione.

L'obiettivo a lungo raggio, in altri termini, è quello di inverare il primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, così come recentemente modificato: far sì che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento europeo, assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Vi sono anche altre motivazioni che spingono verso una radicale riforma della pubblica amministrazione. Anzitutto, occorre superare le vecchie logiche, fortemente radicate nel nostro Paese, improntate al clientelismo e all'assistenzialismo, per cui un impiego massiccio di risorse umane all'interno della pubblica amministrazione è divenuto quasi un surrogato degli ammortizzatori sociali, soprattutto nel Meridione. Occorre, ancora, sradicare il tarlo della corruzione, che sempre più connota l'attività dei pubblici poteri. Trasparenza, efficienza e meritocrazia devono essere le linee guida di una nuova e rinnovata pubblica amministrazione, che sia improntata al buon andamento, come impone la Costituzione stessa, e sia rivolta all'interesse del cittadino, come suggeriscono la logica ed il buon senso. La delega che attribuiamo al Governo con questo provvedimento è sicuramente ampia ed interviene su diverse direttrici, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso del proficuo lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali: dalla Carta della cittadinanza digitale al riordino della disciplina della conferenza dei servizi, dal silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche alla segnalazione certificata di inizio attività, dalle norme in materia di autotutela a quelle in materia di prevenzione della corruzione. Centrali, nell'economia del provvedimento poi le disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici e del personale della pubblica amministrazione, che mirano ad una generale razionalizzazione degli uffici e del personale dell'amministrazione centrale e periferica, con un conseguente riordino di strutture e funzioni. Sul tema, tengo a porre l'attenzione sul nuovo articolo 9 del disegno di legge, che detta norme sull'ordinamento della dirigenza. Il primo comma prevede, in particolare, l'istituzione del ruolo della dirigenza pubblica, articolata in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure di reclutamento improntate non soltanto al merito, ma anche alla formazione e all'aggiornamento continuo. L'obiettivo dichiarato è quello di avere una dirigenza di alto livello professionale, reclutata in modo trasparente e sulla base di criteri meritocratici, che sappia anche e soprattutto adeguarsi ai continui e repentini mutamenti in atto nella società odierna, in modo da evitare il perpetrarsi di quel tipico iato esistente tra pubblica amministrazione e società. La previsione di tre ruoli dirigenziali (dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), della piena mobilità tra gli stessi e dell'eliminazione della distinzione in fasce, unitamente alla previsione di nuove regole di accesso alla dirigenza improntate ad una selezione competitiva e meritocratica, consentono sicuramente di perseguire l'obiettivo di arricchire l'amministrazione di competenze maturate su diversi livelli di Governo. di evitare incarichi a vita, che hanno caratterizzato soprattutto il passato meno recente, è garantita dalla previsione di incarichi di durata triennale, con possibilità di rinnovo, e dalla correlata possibilità di revoca dell'incarico, in presenza di appositi presupposti oggettivi che consentano di evitare un assoggettamento dei dirigenti agli organi elettivi. anche quale antidoto alla corruzione, che la dirigenza pubblica, pur nel rispetto delle competenze e delle specializzazioni acquisite, possa e debba ruotare negli incarichi. In questo contesto si inseriscono anche le norme in materia di segretari comunali e provinciali. In linea con il testo approvato dalla Commissione, ritengo che l'abolizione *tout court* della figura dei segretari sarebbe di per sé priva di logica. Si tratta, infatti, di una figura di primo piano nel quadro dell'attività amministrativa dell'ente locale, chiamata a svolgere funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in relazione alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello Stato, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. L'assenza di tale figura rappresenterebbe un forte *vulnus* rispetto alla necessità di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa e il buon funzionamento degli organi, nell'attuazione del principio di separazione dei poteri di separazione dei poteri tra politica e amministrazione. Si tratta di un ruolo delicato, tecnico e di responsabilità per garantire la correttezza e la legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, la proposta approvata dalla Commissione affari costituzionali (e a proposito voglio ringraziare il Ministro, il Sottosegretario, il relatore e tutti i componenti della Commissione stessa per l'ampia disponibilità e sensibilità mostrate sul tema) stabilisce che l'abolizione della figura del segretario comunale sia adeguatamente bilanciata con la previsione di un obbligo, in tutti gli enti locali, di una figura apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa: direi un punto fermo importante nell'assetto organizzativo dell'ente locale. Ora occorre - mi auguro nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento - fissare ulteriori paletti per garantire la piena autonomia e indipendenza di tale figura apicale, soprattutto nella logica del rafforzamento della funzione di prevenzione della corruzione già assegnata con la legge n. 190 del 2012. Ritengo altresì necessario prevedere criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali per lo svolgimento di tale importante compito, al fine di garantire sempre la terzietà di tale figura professionale nel contemperamento tra l'attuazione dell'indirizzo politico, fissato dal vertice politico dell'ente locale, e il perseguimento della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, nell'interesse dei cittadini e dello Stato stesso. Sono certa che con il contributo di tutto il Parlamento

il relatore, senatore D'Ascola, ha svolto la relazione orale. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

di quelle misure deflattive della popolazione carceraria messe in campo nel tentativo di dare una risposta alla messa in mora da parte della Corte di Giustizia europea ed alle sollecitazioni provenienti dall'allora Capo dello Stato, senatore Napolitano, nel senso di dare sollievo alle condizioni di vita dei detenuti che si pongono decisamente al di sotto degli *standard* dei Paesi civili. A nulla è valso, a mio avviso, il provvedimento di legge approvato, che prevede un risarcimento di sette euro al giorno per ogni giorno di detenzione. Alcune di queste misure sono già legge, come il cosiddetto svuota carceri *bis*, mentre altre sono ancora all'esame delle Commissioni competenti: mi riferisco all'indulto e all'amnistia, provvedimento del quale sono relatore in Commissione giustizia, poi stato sostanzialmente arenato. Sarebbe corretto che la maggioranza chiarisse le proprie determinazioni su questo disegno di legge e che eventualmente lo si scalendarizzasse,

Tuttavia, il disegno di legge sulla riforma della custodia cautelare, al di là della contingenza che l'ha generato, avrebbe potuto essere l'occasione per rimediare a quell'anomalia tutta tipicamente italiana, rappresentata dall'elevata percentuale nella popolazione carceraria di detenuti in attesa di giudizio. L'imputato - non lo dico io, ma la nostra Carta costituzionale - si presume innocente fino alla condanna definitiva. Dunque, la sostanza della carcerazione preventiva - comunque la si voglia definire: custodia cautelare, custodia protettiva o con qualunque altro sinonimo che la fantasia degli uffici legislativi potrà o trovare - non cambia. È ontologicamente ed irrimediabilmente ingiusta, poiché porta necessariamente con sé il rischio di annientare la libertà personale di un uomo, che si presume innocente e che, con percentuali e che, con percentuali che si possono calcolare e non sono insignificanti, sarà dichiarato tale all'esito definitivo del processo. Accettare tale rischio, si badi bene, può essere indubbiamente necessario, ma deve costituire davvero l'*extrema ratio* e l'eccezionalità del ricorso alla carcerazione preventiva dev'essere effettivamente garantita da un sistema di regole chiare e non suscettibili di manipolazioni interpretative. In questo senso, il disegno di legge che stiamo affrontando, sul quale comunque preannuncio comunque un voto favorevole, rappresenta per molti aspetti un'occasione mancata e gli interventi correttivi effettuati nel passaggio tra i rami del Parlamento non hanno certamente risolto le principali criticità di un progetto che resta complessivamente generico, velleitario ed inefficace. Ciò vale anche se è stata opportunamente eliminata la surreale norma dell'originario articolo 3 che, nel riformare il comma 2-*bis* dell'articolo 275 del codice di procedura penale, tra le circostanze impeditive della custodia cautelare, conteneva la previsione - forse sarebbe meglio parlare di divinazione - che, all'esito del giudizio, verosimilmente dopo anni, l'esecuzione della pena sarebbe stata sospesa ai sensi dell'articolo del codice di procedura penale. I passi, però, si sono limitati sostanzialmente a questi; anzi, ricordo che il passaggio alla Camera ha prodotto l'eliminazione di quella parte del disegno di legge che, introducendo un comma 9-*bis* all'articolo 309 del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità per le udienze del tribunale della libertà di un differimento, anche d'ufficio, da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni, quando ciò sia richiesto dalla complessità del caso e del materiale probatorio. Si trattava di un tentativo di rendere la giustizia un po' meno sommaria, soprattutto nei casi in cui il tribunale si trovi ad esaminare ordinanze di migliaia di pagine, coinvolgenti decine di posizioni soggettive, che sono - non dimentichiamolo In questa prospettiva, quindi, ancora una volta sollecito il voto dell'Assemblea sull'emendamento da me presentato per reintrodurre questa possibilità. Per il resto, le criticità rimaste sono tante. Dal punto di vista della tecnica legislativa, infatti, in molti punti si continua a registrare quel florilegio di aggettivi e di formule astratte che, negli anni, hanno sempre dato pessima prova, destinati a scolorire e a perdere di significato nelle prassi degli uffici giudiziari, che le hanno, con l'indubbia capacità dialettica dei nostri giuristi, masticate, digerite ed espulse, riducendole a vuoti simulacri, privi di vita e di significato pratico. Così è avvenuto, infatti, con il passaggio dai «sufficienti» ai «gravi indizi» di colpevolezza richiesti per l'adozione delle misure cautelari. lo ricorderete - e fu salutato, all'epoca, come una rivoluzione, eppure non ha impedito la cosiddetta Tangentopoli, gli abusi della custodia cautelare in funzione di coercizione alla confessione, i suicidi in carcere o alle porte

prima di soffocarsi con una busta di plastica, lasciò, come testimonianza lucida delle pratiche di quegli anni, nelle lettere ai suoi familiari. Ve ne cito un passo e, poiché sono parole scritte da un uomo che, di lì a qualche momento si sarebbe tolto la vita, vorrei pregare i senatori presenti in quest'Aula di ascoltarle con molta attenzione: «Miei carissimi, sto per darvi un nuovo, grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso sopportare più a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna e al rancore dell'opinione pubblica. La mano pesante, squilibrata e ingiusta dei giudici ha fatto il resto. Ci trattano veramente come non-persone, come cani ricacciati ogni volta al canile». E ancora: «La convinzione che mi sono fatto è che i magistrati considerano il carcere nient'altro che uno strumento di lavoro, di tortura psicologica, dove le pratiche possono venire a maturazione, o o ammuffire, indifferentemente, anche se si tratta della pelle della gente. Il carcere non è altro che un serraglio per animali senza testa né anima».

provvedimento oggi in discussione, nella parte in cui aggiunge la locuzione «attuale» a quel «concreto pericolo di fuga» che può giustificare la custodia cautelare, ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale. È evidente, infatti, che un pericolo concreto è certamente anche attuale e che il concetto di attualità si presta alle più estese latitudini interpretative. Anche la stessa idea, che naturalmente è presente nel provvedimento, della custodia domiciliare come misura cautelare ordinaria è realizzata in modo involuto e criptico. Forse la maggioranza se ne vergognava, costruendola infatti, così come l'ha costruita, solo in negativo, con la previsione, introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge, di un nuovo articolo 275, prevede la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere soltanto quando le altre misure cautelari coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Analoghe considerazioni rispetto all'obbligo imposto al giudice, con l'aggiunta di un comma 3-*bis* all'articolo 275 del codice di procedura penale, di indicare, quando applichi la custodia in carcere, le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*. Ma davvero pensate che sia difficile per un giudice motivare e scrivere una motivazione che giustifichi il perché dell'utilizzo della custodia cautelare in carcere e non già di quella alternativa domiciliare? Onorevoli colleghi, chi frequenta per motivi professionali i nostri tribunali ha già avuto modo di vedere provvedimenti applicativi di custodia cautelare in carcere che, ancor prima della riforma che ci accingiamo a varare oggi, già motivano sul tema della necessità della custodia cautelare con argomenti tanto apodittici e pregiudiziali da risultare inattaccabili come dogmi. a mio avviso, sarebbe stato più efficace e lineare, anziché disseminare il percorso motivazionale del giudice di ostacoli puerili e meramente logico‑formali, subordinare il ricorso alla custodia cautelare in carcere esclusivamente al pericolo della commissione di delitti con uso di violenza o contro la persona. Ciò sarebbe stato oltretutto anche più equo in termini di comparizione dei valori in gioco. Soltanto la necessità di proteggere di proteggere il supremo bene della vita e dell'incolumità delle persone può giustificare la massima compressione del bene della libertà personale di un presunto innocente o di un non colpevole (se preferite), rappresentata dalla detenzione inframuraria, con tutto ciò che implica in termini di sofferenza psichica ed esistenziale. Ma ciò implicherebbe un radicale cambio di prospettiva della riforma, che non può essere salvata - mi perdonino i volenterosi colleghi - nemmeno dall'innesto degli emendamenti che operano su una struttura fondamentalmente ed irrimediabilmente errata, per i motivi che mi sono

non ridurrà gli abusi della custodia cautelare, non farà scendere la popolazione carceraria e sarà appunto un'occasione mancata, una delle tante di questa legislatura. tanto alla custodia cautelare, perché, licenziando questo provvedimento di legge, certamente non otteniamo il risultato sperato. Vorrei però rivolgere un appello alla sinistra, alla maggioranza, a questo Governo:

dall'allora Capo dello Stato ed abbiamo ricevuto sollecitazioni dal Papa, per tentare di eliminare questa disumana condizione di vita della popolazione carceraria, determinata essenzialmente dalla sovrappopolazione. Potremmo allora intervenire con il provvedimento di indulto ed amnistia, di cui io e la collega senatrice

soggetti che hanno commesso reati ed avuto condotte di particolare allarme sociale e riducendo al minimo coloro che possono eventualmente beneficiarne. Però non lasciamo un provvedimento così tanto atteso e così tanto sollecitato da varie parti si areni, peraltro con indifferenza. Io allora vi dico: ove mai riteniate che non possa essere approvato, abbiate il coraggio di il coraggio delle vostre idee, il coraggio delle vostre condotte, il coraggio delle vostre azioni.

proposta di legge oggi all'esame di questa Assemblea tratta modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, modifiche alla legge n. 354 del 26 luglio 1975 in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazioni di gravità. La relazione alla proposta di legge, nonostante il titolo altisonante, comincia con il recitare che il problema carcerario in Italia è cronico ed assume dimensioni sempre più preoccupanti, con istituti penitenziari sovraffollati, condizioni detentive sempre meno degne di un Paese civile; un'aggravante della situazione carceraria sotto la pressione di un'ansia di sicurezza, assecondata assecondata talvolta con troppa disinvoltura, che ha prodotto una legislazione emergenziale, solo preoccupata di prevenire e di punire senza preoccuparsi di avere attenzione per le ricadute sanzionatorie complessive. La relazione recita anche che non si tratta soltanto di arginare la piaga del sovraffollamento che da anni caratterizza il nostro sistema carcerario e questa proposta di legge si dà l'obiettivo di affrontare la parte del problema carcerario connessa all'uso tendenziale in chiave preventiva e anche quello di ridurre per legge l'ambito di applicazione della cautela senza incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini e sull'efficienza del processo. Certamente in queste parole immagina di elevare la soglia di applicazione della custodia cautelare ai reati puniti con pena non inferiore a cinque anni senza che venga penalizzata l'esigenza complessiva di sicurezza dei cittadini.

o forse è meglio farlo passare sottobanco, sottotono, alla chetichella, come direbbe qualcuno, nel silenzio generale. E forse la risposta, signora Presidente, è proprio questa. poco clamore su un provvedimento che è legato indissolubilmente ad altri provvedimenti inerenti sempre alla carcerazione preventiva. Questo è l'ennesimo provvedimento, l'ennesimo disegno di legge che nasce ed affonda le proprie radici nella palude del sovraffollamento delle carceri,

carceri. In modo particolare, nei primi mesi di questa legislatura, il tema delle carceri è stato ritenuto il problema principale da affrontare, già con il governo Letta,

Poi c'è stato il decreto-legge del dicembre 2013, che citava nel titolo «riduzione controllata della popolazione carceraria». altro decreto in materia detentiva e non carceraria era quello di sospensione del provvedimento per messa alla prova. La messa alla prova ci è sempre risultata molto simpatica. Tutti questi provvedimenti

Appare evidente - e ne siamo assolutamente convinti - che prima o poi questo Governo e questa maggioranza ci porteranno a un provvedimento clemenziale che forse, una volta per tutte, si avrà il coraggio di chiamare indulto o amnistia.

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Probabilmente al legislatore non sarà parso vero di mettere in condizione l'immigrato clandestino di poter essere ancora più tutelato. l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti in territorio in stato di emergenza. Ne abbiamo parlato in tutte le Commissioni. Abbiamo prodotto fiumi di carta per quanto riguarda l'ILVA e poi andiamo a mettere in condizione questi soggetti di non essere puniti a dovere. lancio di razzi o uso di strumenti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive. Ci siamo sciacquati la bocca tutti, ogni volta che, a fine partita, succedeva qualcosa, sul fatto che probabilmente avremmo dovuto avere leggi più restrittive. Signora Presidente, credo che questo provvedimento rappresenti due fatti, in particolare. Rappresenta una resa incondizionata dello Stato di fronte alla criminalità in un momento in cui lo Stato deve e dovrebbe porre in essere misure per contrastare quei fenomeni di criminalità e mettere in condizioni di essere assolutamente pesante sotto l'aspetto della pena da scontare. In tutte le campagne elettorali c'è sempre qualcuno che ripete fino alla noia che la sicurezza è una cosa molto importante per i cittadini,

(probabilmente uso la parola sbagliata). In un altro intervento che riguardava questi decreti avevo definito il Governo

Signora Presidente, vorrei far presente in quest'Aula che sono giorni oramai che sui giornali della mia amata Regione Liguria non si fa altro che leggere delle aggressioni che subiscono gli agenti della Polizia penitenziaria da parte dei detenuti. L'ultimo, in termini temporali, è avvenuto il 27 marzo scorso nel carcere di Sanremo, dove due agenti sono finiti in ospedale a causa delle percosse ricevute da un detenuto con problemi psichiatrici.

all'interno delle case circondariali della Provincia di Imperia a causa dell'accorpamento con la Regione Piemonte, e l'interrogazione finestra"), con risposta in Commissione, pubblicata il 12 novembre 2014, in cui si denuncia il sovraffollamento delle suddette case circondariali. Ad oggi è stata chiesta un'ispezione ministeriale urgente al DAP da parte delle sigle sindacali della Polizia penitenziaria negli istituiti liguri, dove il personale

detenuti e vorrei sapere come il Governo intenda affrontare questa situazione da considerare inaccettabile per un Paese civile.

bambini e ragazzi. Abbiamo allora tutti condiviso, anche con retorica, la necessità che il Parlamento, il Governo e i vari soggetti istituzionali abbiano a prestare sempre più la massima attenzione ed il massimo sostegno al mondo delle disabilità. Se non che, a meno di un mese dall'inaugurazione di Expo, emergono delle strane sorprese. Non mi riferisco all'iniziativa del Partito Democratico milanese che, per compensare la perdita di tesserati, si permette di pagare il biglietto di ingresso ad Expo

Per le visite scolastiche è stato infatti deciso che, mentre gli insegnanti o gli educatori di sostegno degli studenti disabili hanno l'ingresso gratuito, gli stessi studenti disabili devono invece pagare il biglietto di ingresso. La decisione è doppiamente vergognosa, anche perché la società Expo 2015 ha istituito il "Progetto scuola", un progetto che vorrebbe offrire la possibilità al mondo scolastico di essere protagonista di un percorso didattico e formativo per la diffusione delle corrette abitudini alimentari tra gli studenti, coinvolgendo questi ultimi in esperienze di valore che possano guidarli in scelte alimentari consapevoli.

Con tale interrogazione chiediamo al Governo di adottare un'iniziativa urgente per consentire l'accesso gratuito ad Expo 2015 agli studenti diversamente abili,

intervengano qui tempestivamente, evitando alla decisione ritardi che si aggiungono ai ritardi che stanno - ahimè - caratterizzando negativamente la realizzazione dei padiglioni. Il mondo della scuola, che da settimane sta prenotando le visite scolastiche, non si capacita di questa rozza e inqualificabile decisione. Cerchiamo almeno qui di evitare un'altra figuraccia.

«Una scena da brividi, tra piazza del Bacio e il sottopasso che conduce al Broletto: i poliziotti di quartiere al termine di un'operazione fanno scattare le manette ai polsi di un tunisino e fanno per portarlo in questura. Ma a questo punto succede l'inverosimile: un altro nordafricano vede la scena e, dopo aver chiamato a raccolta altri connazionali, si fionda addosso ai poliziotti tirando fuori la cintura e cercando di colpirli per fargli allentare la presa sul connazionale arrestato. Nel frattempo arrivano gli altri tunisini, e anche loro si fanno sotto con aria minacciosa verso i poliziotti. Ne nasce inevitabilmente un parapiglia, con i poliziotti che cercano e ottengono immediatamente il supporto della squadra volante: una volta sul posto, le forze si riequilibrano e i tunisini sono costretti a dileguarsi non prima di aver cercato di prendere a bottigliate i poliziotti». Un cittadino che ha assistito commenta in questa maniera: «Questi sono convinti che Perugia sia la loro, che sia il loro territorio».

Siamo nella zona di Fontivegge, nei pressi della stazione, una zona che purtroppo si è adeguata, anzi direi abituata al degrado e non adeguata, perché tutto quello che vogliamo è che Perugia non si adegui a questo degrado, anzi il contrario. Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione del Ministro dell'interno riguardo a una simile situazione che si era sviluppata a Varese. Siamo lontani centinaia di chilometri, ma questo significa che ogni città del nostro Paese vive le stesse condizioni di disagio, di degrado e di insicurezza. Invitai il Ministro dell'interno a venire a Varese senza scorta e ad attraversare piazza della Repubblica. Oggi lo invito a passare anche da Perugia, ad attraversare piazza del Bacio, a passare sotto la ferrovia nel sottopasso e ad andare in via del Macello, senza scorta, come un cittadino qualunque, in un'ora serale; si accorgerà del degrado che purtroppo le Forze dell'ordine non riescono più a contenere, perché mancano di strumenti adeguati

In assenza di questi provvedimenti, le nostre città restano preda di queste situazioni. Noi a questo non ci pieghiamo, non si piegano i cittadini di Perugia e invitiamo il Ministro a fare anche questo passaggio. Ogni volta che ci sarà una situazione simile glielo ricorderemo e siamo sicuri che il pellegrinaggio per le città del Paese gli farà solo bene.

L'ACG viene acquistata dal gruppo TeamSystem, che è un'azienda molto solida di Pesaro e che opera prevalentemente nella fascia adriatica. È conosciuta a livello nazionale, ha molte commesse ed è in grado di gestire processi complessi. Per cui,